Signor Sottosegretario, siamo alla trentaduesima, o forse trentacinquesima, questione di fiducia - abbiamo perso anche il conto - e dalle vicende di queste ultime settimane, di questi ultimi giorni è ormai chiaro a tutti che non basteranno uno, dieci, cento decreti milleproroghe a salvare questo Governo e questa maggioranza dalla confusione, dal vuoto, dall'accavallamento di annunci, di proclami, di scelte sbagliate che avete voluto propinare agli italiani in questi ultimi tre anni. Non basterà certamente aver titolato questo decreto, in un'ennesima presa in giro, «proroga di interventi urgenti a sostegno delle imprese e delle famiglie» quando in esso - il Sottosegretario lo sa bene - non troviamo un solo euro aggiuntivo per questi interventi, non una sola risorsa in più, ma solo uno spostamento di poste di bilancio, una diversa allocazione delle risorse stesse, un gioco delle tre carte. Nel nostro Paese, con un milione di persone senza lavoro ed in cassa integrazione, il dato della spesa complessiva per gli ammortizzatori sociali continua ad essere sconcertante. Rispetto al suo PIL, l'Italia spende circa la metà degli altri Paesi europei: meno della Germania, della Francia, del Belgio e siamo agli ultimi posti, insieme alla Grecia e alla Bulgaria. Nelle azioni di aiuto alle famiglie viene confermato anche con questo decreto un panorama desolante, con il Fondo nazionale delle politiche sociali ridotto di un terzo, il Fondo per la famiglia passato a pochi milioni, il Fondo per la non autosufficienza quasi azzerato. Si potrà dire, come dirà certamente qualcuno della maggioranza, che non era questo provvedimento lo strumento, né era questo il momento per affrontare tali questioni. Lo è stato però, come avete dimostrato, come ha dimostrato questa maggioranza, per affrontare invece il problema delle quote-latte, dell'abusivismo edilizio in Campania, dell'aumento degli assessori per il sindaco Alemanno, degli interessi degli oligopoli televisivi, del BancoPosta, degli interessi del sistema bancario. La questione di fondo a cui siamo arrivati, e con cui ora voi della maggioranza siete costretti a confrontarvi, è che il controllo del bilancio pubblico, che pure è cosa importante, poteva e doveva essere affrontato in un modo diverso diverso e sicuramente più equo. Voi avete scelto la strada più facile: avete rinnegato le riforme promesse, non siete stati capaci di investire sul futuro puntando sull'istruzione e la ricerca, l'innovazione. Avete fatto pagare il conto ai lavoratori dipendenti, ai giovani precari, ai piccoli imprenditori, alle famiglie. Tagli alla cieca nei trasferimenti agli enti locali, con la conseguenza di aumenti delle tariffe per i servizi pubblici, le mense scolastiche, i trasporti, l'assistenza agli anziani. E nel frattempo, gli italiani hanno perso in media 1000 euro di reddito a testa, con una recessione che colpisce duramente non solo il Sud, ma anche le più forti Regioni del Nord-Ovest, come la Lombardia ed il Piemonte. Sono questi i dati recenti e drammatici che ci vengono forniti dall'ISTAT. Non vediamo poi spiragli migliori con il federalismo confuso che avete cercato di imporre scavalcando il Parlamento. Si aumenta la tassazione sui fabbricati di artigiani e piccoli imprenditori, si introducono nuove imposte di scopo e di soggiorno e, al contrario, si fanno sconti fiscali, con la cedolare secca, ai grandi proprietari. Soltanto pochi giorni fa il Governo ha fatto finta, finalmente, di accorgersi che bisogna fare qualcosa per la crescita del nostro Paese e ha annunciato l'ennesimo piano per la crescita. È sconcertante, è vergognoso constatare l'inconsistenza avvilente dei provvedimenti proposti, la stupefacente faccia tosta con la quale sono stati presentati, appena mascherati dall'imbarazzo dello stesso Ministro dell'economia, che ha pensato bene di parlare poco e di andarsene prima perché doveva prendere un treno.

Da due anni e mezzo annunciate il piano per il Sud: un piano aggiornato, modificato, ripresentato e mai attuato. Prendiamo purtroppo queste ultime dichiarazioni del Governo per quello che veramente sono, una manovra diversiva, un meschino tentativo di deviare l'attenzione dalle vicende giudiziarie e amorose, diciamo così, del Capo del Governo utilizzando i problemi economici come uno schermo, un ennesimo specchietto per le allodole. Signor Sottosegretario, non basteranno una, dieci, cento questioni di fiducia per mascherare lo stallo politico in cui vi siete impantanati. un Governo senza forze, senza proposte credibili, che cerca una boccata di ossigeno per rianimarsi vendendo al Paese una vecchia telepromozione fatta di chiacchiere e di inganni. È un Governo senza maggioranza. Capiamoci bene, quella maggioranza appiccicaticcia che è stata raccattata, preoccupata soltanto - diciamo la verità fino in fondo - di completare la legislatura, di maturare la pensione ed essere ricandidata se possibile in una postazione sicura, non è una maggioranza. Altro che calciomercato! Il Parlamento è stato ridotto ad un vero e proprio mercato ortofrutticolo, dove i cavoli si possono, certo, comprare a qualsiasi prezzo, si possono anche chiamare con nomi diversi, ma sempre cavoli restano. restano. Il problema vero, il nodo centrale che si nasconde dietro questo scontro violento ed esasperante tra le istituzioni, a cui state costringendo ad assistere non solo gli italiani, ma l'intera comunità internazionale, che ci sta ridendo dietro,

è quello della moralità pubblica come cemento della democrazia, quello della questione morale come condizione essenziale di una convivenza civile, che non si può ridurre soltanto alle vicende di un Capo di Governo che impegna il suo tempo a fuggire dai tribunali e rifuggire nei festini, ma investe invece il rapporto stesso che deve esserci tra il buon ordinamento di una società civile ed il patto stretto tra elettori ed eletti, ed eletti, che impone di essere nelle istituzioni, come ci ricorda la nostra Costituzione, con disciplina e onore. Onore per noi vuol dire l'impegno ad accettare le regole, quelle della giustizia, del fisco, della libertà di informazione, incluso l'obbligo - piaccia o non piaccia - di sottostare alle leggi, come e più di ogni altro normale e privato cittadino! Il problema è tutto qui: e non è poca cosa! La strada per la crescita che il nostro Paese deve inevitabilmente perseguire, se vogliamo dare una speranza ai giovani, alle donne, ai disagi del Sud, al Nord con le sue difficoltà, passa per una grande prova di responsabilità nazionale, che per noi dell'Italia dei Valori è qualcosa di altro rispetto ad un semplice cartello elettorale. Voi, signor Sottosegretario, non avete più la credibilità, non avete la forza né il coraggio di dare una visione e un futuro al nostro Paese. Potevate farlo, ne avevate avuto il mandato, ma chi vi comanda, e che aveva responsabilità di guida di questa maggioranza, ha impiegato il suo tempo diurno e notturno in ben altre faccende.

torni nelle loro mani. Per questo voteremo no alla fiducia. *(FLI)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, i senatori De Angelis, Saia, Menardi, Germontani e Baldassarri hanno esplicitato in Commissione e in Aula le valutazioni di merito rispetto al provvedimento che è stato presentato.

lo hanno fatto anche - in particolare il senatore Baldassarri - attraverso la riproposizione di una proposta complessiva di politica economica. Cito gli interventi dei colleghi perché mi aiutano nella valutazione, nel giudizio e nella sinteticità della riflessione. Aggiungo alcune considerazioni. La prima considerazione è di metodo. Diamo atto ai Presidenti delle due Commissioni, il senatore Azzollini e il senatore Vizzini, di aver concretizzato un metodo positivo di dibattito, di confronto, di ascolto, di apertura al contributo da parte delle opposizioni e delle minoranze per migliorare il testo.

ad una politica economica capace di innescare meccanismi di crescita e di sviluppo tali da accompagnare i segnali di ripresa e consentire a imprese e famiglie di avere fiducia nella prospettiva di disporre di di più risorse e più reddito. Francamente, aver detto no alla proposta cui facevo prima riferimento, ancora una volta ariosa, capace di affrontare con rigore, equilibrio e sostenibilità un punto di sintesi importante tra la lotta agli sprechi, tra la dimensione vera e concreta del rigore all'interno di una manovra importante e significativa caratterizzata da iniziative di crescita, ci porta

La scossa certamente non arriva attraverso un'operazione di revisione costituzionale, peraltro discutibile nel metodo e nell'impostazione, perché quando si mette mano ad articoli importanti e significativi della prima parte della Costituzione non lo si fa a colpi di maggioranza, ma costruendo un consenso all'interno di una proposta più complessiva. Non si dà certo una scossa modificando un articolo della Costituzione, perché comunque, nella migliore delle ipotesi, si determinano effetti di medio e lungo periodo, mentre tutti sappiamo, e basta leggere oggi i quotidiani e lo stesso Ministro lo riconosce con chiarezza, che c'è bisogno di fare di più sul terreno della crescita, della capacità di attivare interventi e iniziative in tal senso. A questo proposito, proprio oggi il ministro Tremonti ci fa sapere che anzitutto bisogno fare di più per quanto riguarda il Mezzogiorno. che il piano per il Sud dovesse determinare chissà quale intervento e chissà quali iniziative: oggi Tremonti ci dice che in sede europea bisogna tentare di negoziare una serie una serie di interventi in relazione alle procedure di appalto e ad eventuali aiuti di Stato, al fine di determinare meccanismi che consentano rapidità d'intervento e che mettano in moto in moto gli investimenti necessari per accompagnare un nuovo intervento nel Mezzogiorno. Questo, francamente, ci pare un ulteriore elemento, seppur di condivisibile riflessione e valutazione, di rinvio rispetto alle questioni ed ai problemi.

abbia bisogno, cioè una sorta di conferenza permanente che metta insieme soggetti istituzionali e sociali, che consenta un'implementazione delle risorse,

nell'ambito di politiche nazionali orientate in tal senso. In attesa ed in mancanza della scossa di carattere economico si continuano però a determinare altri tipi di scosse, che rendono sempre più fragile il tessuto istituzionale, che rendono sempre più difficile il rapporto tra cittadini, politica ed istituzioni, che allargano sempre di più il fossato della credibilità tra cittadini ed istituzioni fino a prefigurare il rischio di una crisi

delle questioni che stiamo tutti affrontando, dello scenario dentro il quale si colloca questo dibattito, fa una sorta di richiamo alla normalità. In fondo è normalità il rapporto tra cittadino e magistratura, e quando il cittadino è Presidente del Consiglio a maggior ragione deve accettare il giudizio; è normalità il rapporto tra Governo e Parlamento. Questa sorta di svolta verso la normalità nei rapporti tra poteri e nei rapporti tra istituzioni può determinare la costruzione di un clima dentro il quale si possa recuperare un confronto alto che superi le contrapposizioni e le lacerazioni, che vada nel segno della condivisione, della responsabilità, della capacità di guardare all'interesse nazionale. È questo che si deve fare, è questo il salto di qualità indispensabile se vogliamo procedere nell'interesse di questo Paese della grande crisi che stiamo attraversando e dell'esigenza di costruire una risposta complessiva all'altezza di tale crisi. Allora, anziché la ricerca affannosa dell'aritmetica parlamentare, anziché questa sorta

di indicare al Paese una prospettiva, una meta e chiamare al senso di responsabilità politico-istituzionale maggioranza ed opposizione in un grande sforzo. In assenza di ciò, se non c'è questa capacità, questa forza e questa volontà, allora si chiuda, si prenda atto del fallimento di un'esperienza, della conclusione di un ciclo e si costruiscano le condizioni, a partire dalla sovranità popolare, per permettere a questo Paese il salto di qualità, per dare la scossa vera, morale, politico-istituzionale di cui ha bisogno.

signor rappresentante del Governo, oggi è un giorno un po' particolare, ed è con un certo imbarazzo che prendo la parola annunciando

6 aprile il Presidente del Consiglio dovrà presentarsi di fronte ai magistrati per essere giudicato. Si tratta di una novità assoluta nella storia del nostro Paese: è la prima volta che il Presidente del Consiglio in carica incappa

Quello che ci domandiamo, però, è dove dobbiamo arrivare, fino a che punto cioè le nostre istituzioni debbano essere umiliate,

come chiunque e, se possibile, con quel maggiore senso di amore per la Patria che dovrebbe avere chi riveste un incarico così importante,

un provvedimento che nega un sostegno reale al Sud e che premia chi in Campania ha commesso abusi edilizi; è un provvedimento che per risolvere i problemi di un manipolo di amministratori capitolini inefficienti ed incapaci fa retromarcia e alza i costi della politica; è un provvedimento che favorisce alcune fondazioni liriche in alcune aree del Paese e ne sfavorisce altre, taglia i fondi per la cultura

Governo, per sostenere ed incentivare le produzioni cinematografiche e continuare a finanziare incentivi fiscali, ha scelto la maniera più semplice: ha scelto di mettere le mani nelle tasche degli italiani

nella speranza che in un comparto così delicato e in crisi un aumento - grazie al prelievo fiscale dell'euro - del 12-15 per cento del prezzo del biglietto del cinema passasse inosservato.

andare a tassare ogni singolo cittadino, avrebbe permesso di finanziare l'intera filiera del comparto cinematografico. L'emendamento che abbiamo presentato sta lì,

non è detto che non si possa seguire da noi: non scegliete sempre la soluzione più facile, quella di mettere, appunto, le mani in tasca ai cittadini, in barba a quanto dite nei dite nei comizi. Noi saremo lì, siamo disponibili a ragionare, e credo che siano disponibili le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali del settore e degli autori. E in proposito, mi viene da domandare: che fine ha fatto il ministro Bondi? Che fine ha fatto l'accordo che il Governo, con Bondi e Tremonti, aveva stretto con le organizzazioni della cultura, gli enti locali e Federculture sul rifinanziamento del

quella furbizia con la quale la Lega aveva portato a casa il finanziamento di 6 milioni di euro destinato solo alle fondazioni liriche aventi sede nelle aree di sua competenza. il ministro Bondi o il ministro Brambilla? Non è, la cultura, un settore strategico per il nostro Paese? Siamo sicuri che l'impoverimento dell'offerta culturale faccia bene all'industria turistica nazionale? Siete sicuri che l'impoverimento dell'offerta culturale faccia bene all'immagine internazionale del nostro Paese? forse, per voi, l'immagine è sufficientemente curata dal Presidente del Consiglio, che oggi campeggia sulle pagine di tutta la stampa mondiale, che tra ieri e oggi ha troneggiato - credo che questo sia il termine giusto nei telegiornali di tutte le televisioni del pianeta: una foto inquietante in prima pagina. Io penso che non sia questa l'immagine che dobbiamo dare di questo Paese.

che, per aumentare e recuperare tre posti in Giunta, entra nella trattativa, nel tritacarne e nella vergogna di aumentare di tre posti anche le Giunte delle altre grandi città, che non

che ne contiene tanti: è un no alla capacità dell'Esecutivo di guidare l'Italia fuori dalle difficoltà in cui versa. È un no a un provvedimento che, per troppi versi, ricorda le finanziarie vecchio stile, quelle dell'assalto alla diligenza. È un no È un no al Governo che aveva risolto tutti i problemi dell'Aquila; è un no al Governo che aveva risolto in via definitiva il problema della "munnezza" a Napoli. È un al Governo che aveva risolto in via definitiva il problema dello sbarco dei clandestini a Lampedusa e sulle nostre coste meridionali. È un no al Governo, colleghi senatori, presieduto da un uomo che non sa governare sé stesso, non sa governare i propri istinti e i propri vizi e, quindi paragmaticamente, non può continuare a governare il nostro Paese.

onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, nella distratta Aula antimeridiana basterebbe rispondere no alla richiesta

poche virtù e nei molti vizi che in questo provvedimento vengono sottolineati. Certo, io sono contento che siano stati trovati i fondi per aiutare i territori colpiti colpiti da calamità. È stato uno sforzo buono e positivo anche da parte del Governo, che ha raccolto le istanze dei territori.

Le proroghe non sono un buon costume, e finiscono per fiaccare davvero quello spirito pedagogico che dovrebbe esservi in ciascuna legge. Ancora di più caratterizza questo provvedimento un grande senso di inappropriatezza, che sta attraversando tutta la società italiana, dentro i suoi grandi sistemi. Sono inappropriati spesso i grandi sistemi sanitari pubblici, che compiono azioni che non devono e fanno male quelle che devono compiere. E così è anche dentro il sistema della legificazione. È curioso, bizzarro e inopportuno un disegno di legge nel quale si può parlare dell'aumento degli assessori della Giunta capitolina e, insieme, anche dei sistemi diagnostici e dei bomboloni sistemi diagnostici e dei bomboloni di GPL nascosti nei giardini. È un provvedimento bizzarro quello in cui si proroga l'inerzia sino all'accidia.

produrre addirittura leggi di sistema, come per Poste italiane o per le banche, in forma di emendamenti. Non credo ci si possa nascondere o trincerare dietro le categorie quali «è sempre stato fatto così» oppure «abbiamo fatto di peggio», come ho sentito talvolta esclamare. Mi sembrano le giustificazioni tipiche di quegli studenti che interrogati rispondono «non c'era sul libro» o «non l'ho trovato». Chi ha l'onere di governare non può fare appello a queste categorie. Credo che, per chi, come me, ma anche per le opposizioni intelligenti, che non fanno il tifo contro il Governo del proprio Paese, anche se sono all'opposizione, deluda il Governo che molto promette e nulla mantiene. Credo che questo modo cattivo di legiferare, che contamina attraverso una modalità impropria anche il Parlamento, finisce con il coincidere con un cattivo modo di governare.

la riforma più urgente sia su come si fanno le leggi, ma credo sia comunque un tema da riprendere e, piuttosto che mandare al macero leggi antiche, che nessuno ricorda più, sarà opportuno rimettere mano presto alle molte contraddizioni che nell'attuale legificazione sono presenti. Non vi immalinconisce davvero il fatto di non riuscire a tradurre minimamente in fatti le molte idee quasi rivoluzionarie che proprio su questo tema avevate proposto?

*(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli membri del Governo, da diversi giorni le notizie prevalenti, o per meglio dire quelle che prevalentemente vengono diffuse e discusse, tendono a far vedere le istituzioni responsabili della guida del Paese vacue ed incapaci, senza valori, obiettivi ed operatività. Non mi interessano i fatti privati, ma gli atti legislativi che si discutono e si approvano per cui non siamo e non ci sentiamo assolutamente indeboliti come qualcuno vorrebbe. Poiché sono convinto che stiamo operando con coscienza e decisione, desidero qui dire ed informare i cittadini sui positivi fatti che questo provvedimento chiamato per semplicità milleproroghe, ma il cui titolo più correttamente è «interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» - contiene, come ora testimonierò.

Sarà così possibile intervenire in Liguria ed in Veneto creando posti di lavoro, economia e sviluppo. E ancora, in merito alle graduatorie del personale docente della scuola,

Proroghiamo l'attività commissariale dell'Agenzia Torino 2006. Finanziamo la gestione governativa della navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como con 2 milioni di euro per l'anno 2011, e consentiamo a a queste gestioni di utilizzare gli avanzi di amministrazione degli anni scorsi. Interveniamo sulle quote latte. La norma sospende fino al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli importi dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte. C'è stato tanto clamore su questo argomento. Noi la riteniamo una misura di buon senso e di giustizia che non ci scandalizza assolutamente.

valore abbiamo in questa disciplina ed è importante, quindi, che sia sostenuta. Interveniamo sul Patto di stabilità, come richiesto e concordato con Regioni, Province e Comuni a dimostrazione della collaborazione vera e produttiva con gli enti locali;

sugli enti parco regionali ove si prevede che i Comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti.

sottolineare che siamo favorevoli alle misure introdotte al riguardo. Sono molti anche i provvedimenti a favore e a riconoscimento del lavoro degli operatori delle forze dell'ordine e della sicurezza a beneficio dei cittadini; i casi degli sbarchi di questi giorni sono emblematici e ringraziamo il ministro Maroni per il pronto intervento. Condividiamo anche le misure di sostegno per il sisma dell'Aquila e dell'Abruzzo; vorrei qui ricordare la solidarietà di tante associazioni e persone che anche dalle nostre Regioni sono andate a prestare il loro aiuto. Richiamo però il collega Lusi per sottolineare che il fatto di aver voluto l'istituzione della Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009, che ha colpito la provincia dell'Aquila e gli altri Comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia, forse è stato una forzatura, un egoismo o egocentrismo e mancanza di sensibilità verso gli altri. parlare inoltre degli interventi sul sistema bancario per mettere in sicurezza le banche dagli attacchi finanziari e, quindi, garantire il risparmio delle famiglie ed assicurare il credito alle imprese, come pure di tanti altri argomenti.

pienamente soddisfatti per quanto fatto ed ottenuto nel segno della fiducia che i cittadini-elettori ci hanno dato, a cui rispondiamo con concretezza, ottenendo un rinnovato sostegno.

*(PD)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, voteremo contro questo provvedimento perché contiene molte misure che non possiamo in alcun modo condividere, perché non contiene alcuni interventi necessari ed urgenti da noi proposti e discussi nelle Commissioni e perché le modalità di esame del provvedimento ed alcune scelte normative tentate o approvate costituiscono la prova che voi, Governo e maggioranza, siete arrivati al capolinea. Non entrerò nel merito delle moltissime misure che compongono il maxiemendamento e delle proposte respinte. Lo hanno già fatto molto bene

alle nostre proposte emendative e a quelle da noi condivise presentate da altri Gruppi, alcune delle quali accolte (ad esempio, quella che restituisce ai precari la tutela dei loro diritti per l'anno in corso), ma anche di un lavoro ad alcune norme impresentabili, come il tentato nuovo condono edilizio o la sottrazione alla giurisdizione della Corte dei conti del *management* della RAI. è stato portato avanti con l'esplicito obiettivo di valorizzare e rendere utile il confronto in sede parlamentare, con la richiesta da noi più volte reiterata di assumere in Aula il testo licenziato dalle Commissioni Commissioni riunite quale base per la decisione che il Governo aveva in qualche modo preannunciato. Abbiamo tenuto ferma questa nostra posizione e diamo volentieri atto a lei, Signor Presidente, e ai presidenti Vizzini ed Azzolini, ai relatori e al Governo, dell'avvenuto rispetto di una regola non scritta, ma da tempo adottata nella prassi parlamentare, secondo la quale quando le Commissioni di merito licenziano testi tanto impegnativi non si possono cambiare le carte in tavola in sede di apposizione della questione di fiducia. Le stesse integrazioni al testo delle Commissioni, al di là del merito delle misure sulle quali abbiamo espresso le nostre posizioni critiche, sono state introdotte nel sostanziale rispetto di tale regola. Non condividiamo, invece, signor Presidente, la tattica dilatoria sin dall'inizio adottata con l'evidente scopo di impedire una lettura piena alla Camera, dove i noti problemi di numeri alla I e alla V Commissione, in particolare, avrebbero certificato già in questa fase l'inesistenza della maggioranza con tutte le immaginabili conseguenze politiche. Queste constatazioni sull'*iter* del decreto non possono però attenuare il giudizio molto critico che abbiamo puntualmente espresso nel corso della discussione. Richiamerò solo alcuni dei principali argomenti, in corrispondenza dei quali si posizionano i sintomi della vostra grave crisi politica. Evidenzio innanzitutto la sostanziale delegificazione della proroga di un numero enorme di termini legislativi (circa 60), già contenuta nel testo originario. Mai ci si era spinti fino a questo punto di forzatura costituzionale: affidare ad un decreto ministeriale, quindi ad una norma regolamentare, il differimento di un termine di legge, calpestando la funzione legislativa e i poteri del Parlamento. Si tratta di una costante di questi tre anni che abbiano più volte denunziato. Parlo poi delle tasse.

per voi che avevate assunto la riduzione delle tasse come dato fondante della vostra politica è un obiettivo clamorosamente disatteso. Non bastava la patrimoniale surrettiziamente introdotta con il federalismo municipale, l'IMU, una imposta sul patrimonio che colpirà artigiani, commercianti, professionisti; né bastava l'aumento delle addizionali sulle imposte, sempre nel nome del federalismo, per rimpinguare le esangue casse dei Comuni italiani. Mancavano alcuni tocchi di fantasia sul sistema tributario italiano in attesa della grande - ripeto - grande riforma. Mi riferisco alla tassa sul cinema: 1 euro ogni biglietto che tutti i giorni pagheranno anche le ragazze, i ragazzi, i pensionati e i disoccupati, quelli che se lo potranno permettere. Non dimentichiamo poi la tassa sulle calamità naturali: un capolavoro di ingegneria tributaria. Su una Regione si abbatteranno terremoti e alluvioni? Alla catastrofe se ne aggiungerà per via legislativa un'altra: l'aumento, al massimo consentito, dei tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e l'aumento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. E se non basterà, dopo l'utilizzo del fondo di protezione civile, bisognerà obbligatoriamente aumentare l'accise sul gasolio. In un colpo solo, signor Presidente, due sacri principi sono abbattuti: il principio di solidarietà da un territorio all'altro del Paese, a fronte di catastrofi naturali, un valore fondativo del nostro Stato; il principio costituzionale della capacità contributiva. *(Applausi dal Gruppo PD).* Se io Stato ti introduco un'imposta, ci deve essere un presupposto, patrimoniale o reddituale che sia, lo dice l'articolo 53 della Costituzione. Qui invece il presupposto è la catastrofe naturale. È incredibile, signor Presidente. ricordo la restituzione delle tasse sospese ai terremotati dell'Aquila (per i quali, pure, sono state introdotte misure utili in Commissione, con l'apporto di maggioranza e opposizione). Il rinvio a novembre del sospeso, necessario anche se non risolutivo, ma senza copertura finanziaria: come si può fare? Come si può aggirare l'articolo 81 della Costituzione? Con un'ordinanza di protezione civile, naturalmente, che è esattamente ciò che prevede questo decreto. Anche in questo caso la fantasia ha oltrepassato ogni limite. Naturalmente, non potevano mancare le quote latte. L'agricoltura italiana è in ginocchio, come ci dicono tutti i giorni le organizzazioni agricole? Niente: non ci sono risorse per interventi, pure proposti con forza da noi Ci sono invece per i truffatori del Nord (per fortuna, dopo le ripetute denunce dei senatori Morando e Giaretta, la Ragioneria ha imposto di ridurre e cambiare quella scandalosa copertura, che Perché si fa l'ennesima norma impresentabile in sfregio al buon senso e alle censure dell'Europa? Perché si pone nel nulla in 24 ore - fatto mai accaduto, signor Presidente una sentenza della Corte costituzionale sui precari della scuola, aggravando il pasticcio nella scuola italiana? Per un solo motivo: perché lo vuole la Lega, l'unico *dominus* del Governo. Nella giornata Nella giornata di ieri, dopo che da diversi giorni si rincorrevano voci in tal senso, il Governo e lei, signor Presidente, avete correttamente investito la Commissione bilancio del tema di primario rilievo del rafforzamento patrimoniale delle banche italiane per via fiscale e bilancistica, in vista dei più rigorosi *stress test* di imminente introduzione con l'accordo europeo cosiddetto Basilea 3. Non ci siamo opposti a derogare alla regola che ho richiamato all'inizio, pur contestando nel merito il contenuto e l'opportunità della norma sull'usura, poi per fortuna stralciata che presentava anche profili penalistici, e quella sulla prescrizione decennale riguardante l'anatocismo, purtroppo confermato. Abbiamo assunto questa responsabilità nei confronti del Paese perché la situazione del sistema creditizio italiano è seria e quando si parla di cose serie noi siamo abituati a fare la nostra parte. Non si può, però, fare a meno di sottolineare che anche qui una delle affermazioni ripetute in questi anni di crisi, «Per fortuna che le banche sono solide» (l'abbiamo sentita tante volte), non era propriamente fondata. Il Governo aveva il dovere di monitorare tale delicatissimo snodo del nostro sistema finanziario ed economico che ne garantisce la solidarietà e la sicurezza e, invece, è costretto ancora una volta ad intervenire perché l'Europa ce lo impone e la Banca e la Banca d'Italia ce lo segnala. Vi è, infine, l'arrembaggio della maggioranza a questo provvedimento con proposte di ogni sorta, come se fosse l'ultima spiaggia, l'ultimo treno prima della conclusione di questa vostra fallimentare esperienza di Governo, sintomo anche che nel Paese sono troppi troppi i fronti aperti e troppi i problemi non risolti, alcuni dei quali li abbiamo segnalati noi, più volte inutilmente, con precise proposte emendative, come l'imminente espulsione di più di 100.000 precari dalla pubblica amministrazione, al netto di quella della scuola e dell'università. Simbolico è il caso dei precari dell'INPS chiamati a smaltire l'enorme mole delle pratiche di cassa integrazione e mobilità e, a loro volta, privati del lavoro *part time* e precario; lo stato di estrema difficoltà degli enti locali, della scuola, dell'università, della cultura, dell'agricoltura e di tanto altro ancora. Aggiungiamo, infine, lo stato comatoso del nostro bilancio pubblico che costringe a disporre coperture scandalose (come quella segnalata dal collega Morando di 100 milioni di euro per il 5 per mille attinti dai crediti d'imposta che, comunque, dovranno essere restituiti alle imprese) e con la certificazione dell'esaurimento ‑ è accaduto anche questo, signor Presidente ‑ a febbraio

e svuotato con le fiducie e con ogni altro mezzo. L'ostentazione di questi anni sull'ordine e la sobrietà degli interventi economici finanziari è risultata vana con il ripetersi dei decreti *omnibus*, più *omnibus* di prima e di sempre. Lo *slogan* di meno tasse per tutti tale è rimasto, uno *slogan* vuoto. La realtà è che le tasse aumentano colpendo anche il cinema; i terremotati e gli alluvionati. La situazione economica e finanziaria e lo stato del nostro bilancio pubblico sono preoccupanti. Il nostro Paese non è fuori dalla crisi e non è purtroppo esente neanche dai rischi finanziari che incombono sull'Europa. Tutto ciò certifica in modo inoppugnabile la vostra crisi politica che, a questo punto, è irreversibile in una fase di grande difficoltà per il nostro Paese di cui siamo seriamente preoccupati. Ruby e dintorni è una in più per il nostro Paese nei confronti delle donne e dei giovani italiani e all'estero. Ecco perché diremo no alla fiducia ed ecco perché è un bene per l'Italia che il Presidente del Consiglio e questo Governo si facciano da parte subito. *(Applausi dai

di ordine quasi costituzionale: dico al senatore Legnini che, peraltro in maniera condivisa, seppur in parte all'interno della Commissione, la questione delle delle proroghe per provvedimento amministrativo è stata sufficientemente sanata, con una previsione di

i decreti ministeriali o i provvedimenti amministrativi verranno dinanzi al Parlamento, alle Commissioni parlamentari competenti. Per quanto riguarda la solidarietà tra territori trova in questo decreto-legge alcune significative conferme, due in particolare: ancora provvidenze, peraltro stabilite insieme, con i colleghi dell'opposizione, verso l'Abruzzo, e altre provvidenze per Regioni che cito proprio perché sono di ogni parte d'Italia. Vi è un emendamento intero che provvede, seppure parzialmente, ad alcuni eventi calamitosi in Liguria, in Campania, in Veneto e a Messina. Questo significa che la solidarietà complessiva verso territori di ogni parte d'Italia è stata confermata: direi, il Centro, il Sud ed il Nord. E questo mi pare inoppugnabile. Così come una serie di istanze che provengono dal mondo dell'editoria, televisiva locale e di giornali, e dello spettacolo hanno trovato in questo decreto delle significative appostazioni di bilancio; certo, meno di quelle richieste ma, come ha detto il senatore Legnini, in un momento di crisi bisogna fare delle scelte e queste sono le scelte che sono state fatte. In ogni caso, questo provvedimento, con il lavoro parlamentare, ha dato delle risposte concrete sia ai problemi dell'editoria, che dell'emittenza locale, che dello spettacolo. Peraltro, nella versione finale, vi è un allargamento a settori importanti, che sono stati oggetto anche di attenzione della stampa, come le fondazioni lirico-sinfoniche.

Il precariato probabilmente proviene da un'idea della sinistra di inserimento dei lavoratori senza concorsi, senza osservanza dei precetti costituzionali. Potrei Potrei darvi degli esempi concreti. Quando vorrete, ragioneremo sul concreto, come nostro solito, nelle Commissioni. Stiamo cercando di eliminare questa situazione, che toglie dignità ai lavoratori: cerchiamo pertanto, lentamente ma inesorabilmente, di di tagliare con quel modo di reclutamento e di iniziare con un modo di reclutamento che rispetti insieme la dignità del lavoro e il merito e non penalizzi coloro che non noi ma altri hanno reso precari. altri hanno reso precari. Noi cerchiamo lentamente di riassorbirli, nel rispetto della dignità, e introducendo peraltro dei criteri di merito. Per quel che riguarda le banche e i fondi, senatore Legnini, credo che il Governo stia monitorando

sia la questione dei cosiddetti *stress test* delle banche, che entro questa primavera saranno fatti in ambito europeo, sia il problema dell'adeguamento dei *ratios* patrimoniali alle

possiamo rimanere di opinioni diverse, ma cominciamo ad affrontare la questione. D'altra parte, va riconosciuto ai colleghi dell'opposizione che, nell'ambito della procedura parlamentare, di cui dirò fra un momento, essi hanno consentito che tale inserito in questo provvedimento, riconoscendone l'urgenza. È un dato che è stato condiviso, fermo restando il nostro giudizio di merito. Lo stesso discorso vale per l'allineamento delle aliquote fiscali dei fondi di investimento, che altro non è che un tentativo di dare respiro al risparmio azionario in Italia e di contribuire alla soluzione di quel problema che molto correttamente ha posto il senatore Morando, cioè il nuovo tentativo di allocazione delle risorse per favorire lo sviluppo, mentre tale sviluppo comincia a profilarsi all'orizzonte dell'economia italiana. Ed è chiaro che il sostegno dell'investimento azionario ne è una delle componenti essenziali. Mi pare quindi che

Innanzitutto, credo che abbiamo scritto tutti insieme - e lo rivendico, spero con i colleghi dell'opposizione - una bella pagina parlamentare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, avremmo voluto che questo provvedimento avesse contenuti più coerenti rispetto ad un percorso, soprattutto per quanto riguarda le questioni economiche, che insieme ad altri colleghi del Gruppo avevamo prospettato. Tuttavia, così come spiegato dal presidente Viespoli, questo provvedimento normativo è di carattere urgente: basti pensare alla necessità di mettere in sicurezza le banche. banche. Ritenendo che la corresponsabilità nel guardare all'interesse nazionale, essendo il voto carico di ragioni istituzionali, non ci debba portare a farci carico di un segnale negativo, per questo aspetto, dichiaro di non partecipare al voto. presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.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

Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia,

Vita,

Di Giovan Paolo, Di

Esposito; Fantetti,

n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia***

Signora Presidente, colleghi, il provvedimento che stiamo per esaminare proroga per i primi sei mesi dell'anno le autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni internazionali. L'entità complessiva degli stanziamenti ammonta a 754 milioni e 300.000 euro ed è sostanzialmente in linea con lo stesso stanziamento del secondo semestre dell'anno scorso.

mentre i restanti 692 milioni e 346.000 euro sono destinati a coprire le spese per missioni militari, confermando il rapporto che nel corso di questi anni si è venuto a definire tra le due componenti, cioè le missioni militari e le altre attività che il nostro Governo ha affidato alle nostre truppe. Di questo però parlerò Vorrei osservare preliminarmente che il provvedimento conferma quella che abbiamo chiamato una linea multilateralista, per cui l'Italia assicura il nostro Parlamento ha già ratificato e condiviso e su cui anche l'opinione pubblica nazionale ha espresso più volte, in situazioni qualche volta spiacevoli, qualche volta positive, il proprio consenso.

confermandosi uno dei principali strumenti di politica estera, che tuttora garantisce la presenza nei principali fori internazionali di decisione strategica. una scelta di fondo della nostra politica estera quella di avere un approccio complementare fra la dimensione militare e la dimensione civile: sono due componenti che avanzano di pari passo e che ci permettono di essere contemporaneamente impiegati non solo nelle operazioni di sicurezza ma anche nel settore umanitario. Abbiamo un compito molteplice in queste aree, non solo di assistenza umanitaria ma anche di sostegno alle amministrazioni locali,

Questo, come premessa generale. Passando ai profili di competenza della Commissione affari esteri, vorrei innanzitutto mettere in rilievo l'Afghanistan, dove sarà operativo nel primo semestre dell'anno un contingente di 4.350 uomini. Sappiamo quanto la situazione politico-istituzionale dell'Afghanistan sia degradata e qual è stato purtroppo il prezzo che abbiamo pagato sul campo. La nuova strategia del generale Petraeus punta

si sarà dimostrato vincente: però fin d'ora sembra necessario affiancarvi una forte iniziativa politica che consolidi il consenso fra gli alleati. quanto riguarda l'Afghanistan. In favore del Libano il provvedimento prevede alcuni interventi sul versante multilaterale a sostegno del programma delle Nazioni Unite per la realizzazione di attività di *capacity* *building* rivolte alle amministrazioni locali e dispone l'erogazione di un contributo di circa 800.000 euro al tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, attualmente al centro di un il nostro contingente non ha soltanto una missione militare da svolgere ma soprattutto o in gran parte una missione di diffusione e Per quanto riguarda il quadro iracheno sono previsti interventi nel settore sanitario, nel settore sanitario, inclusi la formazione e l'addestramento, e in quello della gestione delle acque per il miglioramento della vita nei villaggi. È un problema che anche l'ONU ha sollevato, e il nostro contingente ha delle istruzioni piuttosto precise al riguardo. al riguardo. Si prevede inoltre il finanziamento del programma avviato in favore delle vittime delle torture e delle persecuzioni religiose (ancora una complementarità con la presenza militare). Quanto all'Africa subsahariana, si segnala l'autorizzazione di spesa di 2 milioni e 750.000 euro ad integrazione degli stanziamenti già assegnati anche in riferimento al contrasto della pratica - di cui ci siamo già occupati - delle mutilazioni genitali femminili. Venendo ai processi di stabilizzazione nei Balcani occidentali, il ruolo italiano è stato e continua ad essere molto rilevante e si riflette in una significativa presenza delle Forze armate e di polizia

In tale prospettiva, anche per il prossimo semestre si conferma il dispiegamento di un contingente di 650 unità, in continuità con quanto previsto per il secondo semestre del 2010, anche in un'ottica di protezione dei luoghi di culto della chiesa serbo-ortodossa. Un contributo è stanziato per il finanziamento delle attività dell'Iniziativa adriatico-ionica, la cui presidenza di turno è attualmente affidata all'Italia.

delle convenzioni tra il mondo produttivo della sponda ionica e quello del Mediterraneo, segnatamente la zona che va da Ancona in giù.

Infine, nel I Capo del provvedimento, sono state introdotte dalla Camera una serie di disposizioni tecnico-amministrative per garantire l'effettiva spendibilità, senza troppi legami

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci ritroviamo ancora nella cadenza semestrale, ormai in uso da diverso tempo, seppure con qualche eccezione verificatasi in passato, esaminare, come ricordava il collega Bettamio, il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, come ormai comunemente viene definito. In questa circostanza si ha qualche volta la tentazione di limitarsi all'indicazione di alcuni elementi fondamentali, cosa che comunque chi parla farà nel prosieguo del breve intervento a titolo di relazione, dimenticando che quanto viene prorogato, o ciò di cui in questa circostanza si parla, è spesso oggetto di discussioni e di richieste da parte di colleghi parlamentari dei due rami del Parlamento per la verifica costante degli orientamenti del nostro Paese, segnatamente del Governo, in ordine alla politica estera che

sbagliato attardarsi in polemiche rinviando gli eventuali approfondimenti sulle diverse missioni in cui il nostro Paese è impegnato (che sono molte, come si desume dall'elenco contenuto nell'articolo 4 del decreto‑legge in conversione), e che queste occasioni, cadenzate con tempi sostanzialmente fissi, possano invece diventare l'occasione, appunto, per svolgere quegli approfondimenti e quei dibattiti che tante volte si richiedono e che poi, nelle occasioni in cui sarebbero istituzionalmente previsti, non vengono svolti, oppure si riducono ad alcune parole e clausole di stile.

di strumento legislativo che definisca in maniera sostanzialmente puntuale, ma in qualche modo anche definitiva, gli aspetti salienti della disciplina contenuta in questi decreti, ormai a cadenza tendenzialmente semestrale, ritenendo che queste circostanze potrebbero essere superate da un intervento di questo genere. Personalmente non sono contrario a questa impostazione, ma credo che per molti versi alcuni aspetti - e segnatamente quelli di natura finanziaria - sarebbero sempre e comunque da ripetersi con certe cadenze temporali. In effetti, c'è da domandarsi se possa essere opportuno, in accoglimento di queste richieste, prevedere in qualche modo un quadro di riferimento normativo

puntuale del provvedimento, e specificamente all'articolo 4, dopo le note che sono state riferite dal collega Bettamio riguardo agli interventi di natura civile ed alla parte relativa alla cooperazione

o dell'Unione europea, l'Italia costituisce il quarto contributore in termini di unità e di partecipazione a livello militare. Questo impegno per il nostro Paese, massiccio,

stanziamenti magari più contenuti, i quali però necessitavano poi di un intervento di completamento da parte del bilancio ordinario della Difesa, andando così fortemente ad incidere su quelle contrazioni di cui spesso si parla in ordine, appunto, alle spese della Difesa. alcune edizioni dei decreti a questa parte, infatti, la spesa in essi indicata è quella omnicomprensiva, che non riguarda soltanto le spese dirette e vive, ma anche quelle che che comportano le attività di manutenzione, di ripristino, di consunzione dei mezzi e quant'altro, vale a dire quella sorta di spese indirette che comunque incidono in maniera non indifferente sul totale dell'impegno economico. allora che sia un elemento positivo, non solo di chiarezza e trasparenza per l'esame da parte del Parlamento, aver indicati tutti gli oneri economici e averli riferiti esplicitamente al Fondo previsto nella legge finanziaria per le missioni internazionali, e non farne gravare più una parte sul bilancio ordinario della Difesa, che già ha i suoi problemi.

pluriennale anche dei nostri contingenti. Ma non vanno misconosciute e dimenticate le altre missioni, che dobbiamo sempre ricordare, in tanti altri scenari del mondo, e che sono

per l'incidenza in termini di impegno da parte delle Forze armate italiane, le missioni per il contrasto della pirateria nell'Oceano Indiano al largo delle

da interventi di ricostruzione del quadro istituzionale e di governo. Così come credo debba essere sottolineato quanto indicato al al comma 30 dell'articolo 4, cioè uno stanziamento specifico in ordine al mantenimento del dispositivo operativo dell'Agenzia di informazione e sicurezza estera del nostro Paese per il rafforzamento del quadro di *intelligence*, che spesso giustamente si invoca in ordine sia alla protezione dei contingenti italiani all'estero, sia in generale per la

ambiti internazionali. Al comma 32 è previsto un intervento che in realtà si riferisce ad una situazione diversa, e che autorizza il Governo alla cessione di quattro unità navali della Guardia costiera - Capitaneria di porto al Governo della Repubblica di Panama nel quadro delle intese che con quel Governo sono intervenute. L'articolo 5 del provvedimento reitera ancora una volta le varie disposizioni in ordine al trattamento del personale impegnato nelle varie missioni ed alle competenze che vengono riconosciute a seconda delle diverse situazioni e circostanze. In questo quadro, la Camera dei deputati ha inserito alcuni emendamenti, in parte approvati in Commissione e altri approvati in Aula, e in particolare una disposizione che intervenendo in forma modificativa sull'articolo 884, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, ha effettivamente di lacuna riguardo all'applicazione retroattiva per una disposizione riguardante l'aspettativa

manifestati in anni recenti: si tratta dei casi riferiti allo stato di prigionia di nostri militari piuttosto che alla condizione di disperso. Ritengo sia stato utile questo inserimento e questo completamento attraverso l'emendamento approvato dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, così come l'intervento che si riferisce a una questione spesso oggetto di importanti discussioni e che è intervenuta, in forma modificativa, sull'articolo 603, commi 1 e 2, dello stesso codice dell'ordinamento militare, militare, che ormai raggruppa tutte le disposizioni in materia di difesa e che è entrato in vigore l'ottobre scorso. In questo caso ci si riferisce al riconoscimento della causa di servizio per i previsti indennizzi al personale militare, e anche civile, che abbia contratto infermità o patologie di natura tumorale a seguito della partecipazione a missioni o alla presenza in luoghi e siti dove si riscontrino particolari forme di esposizione a rischio. Questa norma intende in qualche modo semplificare

e, in particolare, anche quelle che hanno introdotto, seppur temporaneamente, per ora, una scriminante speciale, una causa di giustificazione speciale e norme particolari in materia procedimentale per quanto riguarda il sequestro dei mezzi, le perizie dei mezzi militari coinvolti in attentati o, comunque, in incidenti di natura dolosa da parte delle controparti e degli

di un nuovo codice penale militare, definito delle missioni internazionali, nel segno di quanto più volte i due rami del Parlamento, proprio in occasione dell'esame dei decreti come quello oggi, hanno chiesto a gran voce: appunto, la previsione di norme penali militari specifiche che, in qualche modo, conciliassero la diversa e non più tradizionale natura degli interventi militari italiani nei contesti attuali, che difficilmente possono essere ricompresi nella disciplina penale militare di pace, così come in quella penale militare di guerra che, peraltro, opportunamente il Governo Berlusconi aveva invece reintrodotto per le due missioni dell'Afghanistan e dell'Iraq.

affettuoso proprio a coloro di cui in questa circostanza più ci occupiamo, perché non è mai da dimenticarsi che questi provvedimenti si riferiscono a coloro che hanno a mente la bandiera italiana, il senso dell'onore e l'importanza

*(PD)*. Signora Presidente, si ripete spesso, e giustamente, che la discussione sul provvedimento che rinnova le missioni internazionali rappresenta un momento centrale del confronto parlamentare sulla nostra politica estera. Ne hanno parlato anche i relatori nei loro interventi. In realtà, ciò è vero solo parzialmente, poiché, quando si discute dei decreti-legge di proroga, in via generale ci si limita a stabilire le risorse da destinare alle varie missioni internazionali oltre a fissare norme di carattere organizzativo, ovvero soffermare la nostra analisi ed attenzione sulla missione che in quel particolare momento desta grande preoccupazione nell'opinione pubblica. È necessario fare un passo in avanti, uscendo dalla prassi della decretazione d'urgenza per addivenire alla definizione di un'iniziativa parlamentare in grado, anche con la collaborazione attiva del Governo, di fissare il quadro per una nuova organica disciplina giuridica delle missioni internazionali. L'orientamento espresso dal relatore, senatore Gamba, credo possa essere un utile terreno di confronto. Si tratta in buona sostanza di marcare il perimetro nel quale consentire al Parlamento e allo stesso Governo di realizzare un confronto di merito, sia sull'impegno complessivo del nostro Paese nelle aree di crisi e nel rispetto dei nostri impegni internazionali, sia di provvedere ad una disamina attenta di ogni singolo particolare intervento. Situazioni complesse, quali quelle dell'Afghanistan, dei Balcani e del Libano necessitano di valutazioni ed analisi ben più approfondite di quelle che offre la procedura fin qui seguita. L'obiettivo finale è di ridare al Parlamento l'opportunità di discutere con la necessaria profondità ciò che all'estero siamo impegnati a fare con i nostri contingenti militari o con le organizzazioni non governative, insomma con la nostra politica estera. Tra l'altro, proprio gli improvvisi rivolgimenti di quest'ultimo periodo e il corso delle vicende in Tunisia e in Egitto, ma anche in Kosovo, dove esiste il rischio che la crisi tra il *premier* Berisha e il capo dell'opposizione Rama possa degenerare, mostrano chiaramente come ci sia costante bisogno di sedi appropriate di confronto, non dovendosi l'azione parlamentare limitare alle pur doverose comunicazioni del Governo alle Camere sulle eventuali situazioni di crisi che di volta in volta si possono presentare. Inoltre, la procedura fin qui seguita impedisce una soddisfacente valutazione dei diversi contesti nei quali l'Italia è chiamata ad operare. Sembra che gli impegni nelle missioni vengano decisi non nel quadro di una politica complessiva, ma quasi esclusivamente da motivazioni di cassa. Ad esempio, si intende aumentare il numero dei militari impegnati nel nostro contingente in Afghanistan, ma non risulta del tutto chiara la strategia sottesa ad una tale rilevante decisione, che si accompagna ad una riduzione dei nostri contingenti in Libano e nei Balcani, senza che sia offerta una precisa valutazione di merito di quelle specifiche situazioni. È del tutto evidente che la nostra contiguità con l'area balcanica meriterebbe da sola un dibattito, che non può essere sostituito da un sì o un no su un articolo del decreto-legge di proroga. Ricordo a tutti voi che la presenza wahabita in Bosnia è motivo di preoccupazione per le stesse componenti musulmane moderate, e dovrebbe esserlo anche per noi. In ogni caso, la riduzione dell'impegno militare andrebbe almeno compensata da una più accentuata iniziativa di cooperazione, mettendo a disposizione più risorse economiche e un'attenzione politico-diplomatica più decisa. E qui veniamo ad un altro punto critico. La parte relativa agli interventi di cooperazione e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione rappresenta circa il 3,6 per cento dei 754 milioni di euro stanziati per la prima metà del 2011.

Rispetto all'ultimo decreto le risorse per interventi di cooperazione allo sviluppo subiscono una contrazione pari a circa il 10 per cento. Anche includendo nella quota cooperazione iniziative assolutamente strategiche ed importanti come l'iniziativa adriatico-ionica e l'INCE, credo che il piatto pianga. Non c'è bisogno di ricordare che gli interventi di cooperazione allo sviluppo costituiscono un elemento fondamentale e imprescindibile per la riuscita delle operazioni nelle quali il nostro Paese si trova impegnato, posto che sull'efficacia degli interventi incide non solo l'elemento militare, ma certo, e soprattutto, anche quello civile. Lo stesso generale McChrystal, signora Presidente, ex comandante delle truppe Usa in Afghanistan, ha più volte sostenuto, anche in documenti ufficiali, che senza l'azione civile i problemi di quel Paese resteranno irrisolti. In futuro, quindi, è auspicabile una risposta positiva da parte dello stesso nostro Governo.

La forte richiesta di democrazia nelle regioni del Nord-Africa e della Mezzaluna fertile è accolta con soddisfazione da tutti, anche se desta preoccupazione la possibilità che movimenti violenti possano compromettere la sicurezza del nostro Paese. Queste considerazioni generali relative alle vicende in aree vicine rivalutano le decisioni assunte negli anni passati dal nostro Paese in merito alla partecipazione alle missioni E il decreto di proroga, al di là della sua funzione finanziaria, diviene l'occasione per richiamare, da un lato, le caratteristiche di quelle missioni e per valutare dall'altro, se ancora sussista la necessità della loro prosecuzione. Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia le caratteristiche delle missioni, la partecipazione nazionale risponde a impegni che il Paese ha assunto negli organismi internazionali di cui fa parte. L'ONU, la NATO, l'Unione europea, l'OSCE, sono organizzazioni nelle quali l'Italia svolge un ruolo importante, anche grazie alla sua partecipazione alle missioni. Questa partecipazione, inoltre, trova esplicito riferimento nella Costituzione, che all'articolo 11 prevede anche la possibilità di rinunciare a prerogative nazionali a favore degli organismi internazionali, che perseguono obiettivi di pacificazione e stabilizzazione nelle aree di crisi. Nelle operazioni per la pace, infine, la componente militare è quella a cui è affidata la fase iniziale di emergenza, propedeutica alle fasi di ricostruzione e di sviluppo a cui sono preposte altre componenti delle missioni. Proprio perché legato a contesti spesso non completamente pacificati, l'impegno delle forze nazionali ha assunto talvolta caratteri conflittuali, determinati sempre comunque dall'attività e dalle violenze di chi si oppone al processo di stabilizzazione democratica.

avendo ben presente che la legittimazione delle missioni deriva dal tipo e dall'importanza dell'organizzazione internazionale che ne dispone l'avvio e dal livello di condivisione delle decisioni. Ebbene, le operazioni a cui partecipa l'Italia sono state tutte avviate su specifico mandato dell'ONU, ossia in una cornice di massima legittimazione. Per quanto attiene al secondo aspetto, ossia alle valutazioni relative alla prosecuzione dell'impegno nazionale nei diversi teatri operativi, non sono emerse indicazioni che inducano a ritenere completamente raggiunti, in quei teatri, gli obiettivi di stabilizzazione auspicati. In Libano, la situazione politica e le milizie in campo impongono una continua azione equilibratrice delle Forze della missione UNIFIL. Al nostro Paese, che tanto ha fatto negli anni passati per evitare che le storiche tensioni dell'area sfociassero in conflitti pericolosi, compete ancora l'impegno di promuovere tutte le iniziative politiche per scongiurare comportamenti ed atteggiamenti pericolosi. Per quanto attiene al Kosovo, lascia perplessi l'accelerazione della NATO per il disimpegno dalla regione. I timori manifestati a più riprese dalla minoranza serba del Paese, la continua minaccia ai luoghi di culto della religione serbo-ortodossa e la scarsa integrazione tra le diverse etnie impongono di valutare con grande attenzione ogni ulteriore riduzione del contingente italiano, già destinato a contrarsi fino a sole 600 unità.

maggiore presenza di forze sul terreno, ma anche maggiore attenzione al sostegno alla popolazione; accelerazione della formazione delle forze di sicurezza locali, condizione indispensabile per l'«afghanizzazione» della crisi, ma anche massima cura nell'evitare vittime civili; lotta alla corruzione degli apparati afgani, ma anche accentuazione dell'azione politica della comunità internazionale e coinvolgimento dei Paesi moderate e responsabili. Concludo il mio intervento, signora Presidente, con due annotazioni. La prima è relativa alle modalità con le quali il Parlamento affronta l'esame delle missioni internazionali. Il Senato dedica oggi solo poche ore ad un argomento che meriterebbe ben altri approfondimenti e ben altra partecipazione parlamentare, considerato il rilievo che riveste per la politica estera del Paese. Sarebbe necessario prevedere ampie discussioni sulla tematica, così come chiedeva l'ordine del giorno firmato da tutti i Gruppi parlamentari ed accolto dal Governo nel 2009. La seconda annotazione è relativa a coloro che sono l'espressione di questo impegno italiano nelle missioni per la pace: gli uomini e le donne in uniforme delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, nonché gli operatori civili della cooperazione italiana.

pagando di persona, spesso tragicamente, l'attaccamento alla Nazione e l'amore verso la funzione di pacificazione svolta. La sua attività operativa

la sottostima dell'impegno per la pace che svolge ogni giorno, sol perché opera, come fanno i militari, con le armi. Bisognerebbe ricordare a quelle persone che esistono situazioni nelle quali solo la componente militare può integrare i principi di solidarietà, generosità e sostegno di chi soffre con le esigenze di sicurezza

gli studiosi di storia del pensiero costituzionale pongono la funzione informativa come fondamento delle istituzioni parlamentari. Essa dovrebbe, infatti, essere la premessa essenziale di ogni potere legislativo, dato che la legge è l'espressione della capacità di normare decisioni e comportamenti; la funzione informativa è dunque la premessa di ogni democrazia. Sta poi ad ogni Parlamento e ad ogni parlamentare trasferire l'informazione ai cittadini e regolare la sua attività legislativa a partire da questa. Ugualmente l'impianto democratico dell'Europa è in grado di fornire le informazioni sulle principali questioni nelle quali gli Stati dell'Unione europea sono impegnati. Quindi, per affrontare correttamente il tema del conflitto in Afghanistan e quello della nostra missione in quel Paese, voglio porre come esaustiva premessa (evidentemente non ideologica) il contenuto della risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre dell'anno scorso su una nuova strategia per l'Afghanistan. Il documento, infatti, molto dettagliato ed esplicito nelle sue diverse parti considera come oggettivi elementi che è bene diventino di pubblica condivisione. Quindi, la sua lettura in Aula mi sembra importante.

Il quadro, però, è fosco. Nella risoluzione si dichiara - citerò molto spesso le parole precise virgolettate che «né la coalizione di forze internazionali risulta capace di sconfiggere i talebani, né al momento il movimento insurrezionale e talebano risulta capace di prevalere sulle forze militare e quindi» sempre la risoluzione «non si intravede alcuna conclusione certa in Afghanistan». Vengono riportate le considerazioni del generale McChrystal, il quale nel 2009 affermava di «non ravvisare segnali di una forte presenza di Al Qaeda in Afghanistan» e e che «alti funzionari americani confermano che Al Qaeda è oggi scarsamente presente in Afghanistan». Si considera che «le condizioni di vita e di sicurezza in quel Paese si sono deteriorate, erodendo il consenso popolare di cui godeva a un certo punto la presenza della coalizione e

l'impossibilità di una soluzione militare in Afghanistan e che gli Stati Uniti hanno dichiarato che inizieranno a ritirare le loro truppe dall'estate 2011, mentre altri Paesi o l'hanno fatto o stanno mettendo a punto piani per procedere in tal senso». procedere in tal senso». Il Parlamento europeo è altresì consapevole della necessità «di rispettare gli impegni assunti con il Governo afgano per migliorare la sicurezza, la *governance* e le opportunità economiche per i cittadini di quel Paese. Si constata però che, nonostante i miglioramenti realizzati dopo la caduta del regime dei talebani, si è registrato un peggioramento della situazione per quanto riguarda la libertà di espressione e di stampa, così come sono state registrate irregolarità nei procedimenti giudiziari del Paese, non rispettando le norme internazionali in materia, e si continuano ad eseguire condanne a morte». Il Parlamento europeo «riconosce la percezione diffusa secondo cui la corruzione del Governo afgano è la sola responsabile della mancata fornitura di servizi essenziali ai cittadini e ritiene che la lotta contro la corruzione dovrebbe costituire la pietra angolare del processo di pace Tra l'altro, dei 40 miliardi di dollari USA destinati agli aiuti in quel Paese, solo 6 miliardi sono pervenuti al Governo afgano tra il 2002 e il 2009, mentre gli altri 34 miliardi sono passati attraverso organizzazioni internazionali, banche, appaltatori internazionali, ONG, senza raggiungere i beneficiari destinatari, cioè il popolo afgano. Il Parlamento europeo si dichiara costernato - mi sembra di una gravità assoluta che questa ufficiale - per il fatto che il denaro proveniente da attività di protezione a tutti i livelli della catena di approvvigionamento militare costituisca la più significativa fonte di finanziamento dei ribelli, come riconosciuto nel 2009 dalla stessa Clinton, ed è altrettanto costernato dal fatto che allo stesso modo i finanziamenti ISAF possano finire nelle mani dei ribelli, dato che analoga è la logistica militare tra Stati Uniti, NATO e ISAF. Il Parlamento europeo ritiene che l'impostazione militare del passato non abbia dato i risultati auspicati e riconosce che che «l'unica soluzione possibile è di natura politica e ritiene che dovrebbe comprendere i negoziati, da svolgersi eventualmente sullo sfondo di un cessate il fuoco, con i talebani ed altre formazioni combattenti» che evidentemente devono fornire garanzie «nonché con altri esponenti politici del Paese disposti a formare un Governo di unità nazionale che possa mettere fine alla guerra civile che sconvolge il Paese da quasi 30 anni e garantire il pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali». Oltre alla risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2010 di cui ho dato lettura ampia, voglio qui riportare alcune considerazioni pubblicate sul numero zero, arrivato ad alcuni di noi,

Qui si afferma che dopo otto anni di operazioni ISAF la sicurezza in Afghanistan è peggiorata, che in realtà «il nemico che ISAF e *Enduring Freedom* ritengono ancora attivo di fronte alla potenza delle forze occidentali, è numericamente irrilevante e qualitativamente nullo a fronte delle forze NATO presenti». Di seguito si può leggere che nell'Afghanistan odierno, la Costituzione, scritta dagli occidentali, lega il potere laico al Corano, le truppe di polizia dell'esercito non sono viste come risorse nazionali, ma come esecutori materiali di abusi, crimini e corruzione gestiti da un centro che

Concludendo ho voluto riferire all'Aula considerazioni molto significative e, ribadisco, non ideologiche, date le fonti, che forniscono un quadro assolutamente preoccupante dello stato del conflitto afgano. Lo faccio poiché oggi parliamo di un rifinanziamento significativo dal punto di vista economico per altri sei mesi della nostra missione. È per l'evidenza e l'autorevolezza delle fonti che ho qui citato che ho sottoscritto convintamene l'ordine del giorno G102 presentato dal senatore Di Giovan Paolo con il quale si impegna il Governo a promuovere un confronto con i Paesi

al reiterarsi di questo decreto legge lo si evince chiaramente nel titolo un po' ipocrita, che assommando il 4 per cento delle spese per la cooperazione allo sviluppo al 96 per cento delle spese per le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, ogni sei mesi propone la copertura economica di missioni che, pur legalmente munite, non godono né di un quadro giuridico costituzionale né di un quadro legislativo ordinario, nonostante da due anni e 300 giorni circa siano depositati disegni di legge costituzionali e ordinari in materia. Meno retorica patriottarda e più spirito patriottico vero imporrebbero questa scelta al servizio dei nostri militari, dei nostri cooperanti per la pace, dei nostri diplomatici e funzionari. Su questo verte la nostra critica, sull'incerto confine tra spesa militare e cooperazione, sulla situazione di ognuna delle oltre 30 missioni militari e sulla strategia di realizzazione degli scopi e, certo, anche sull'*exit strategy* in Afghanstan che, assieme ai Balcani e al Libano, rappresenta uno dei punti nodali dell'impegno italiano. Su questo ci sono tre ordini del giorno di cui uno è la copia dell'ordine del giorno approvato all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari in Commissione 14a. Mi aspetto la loro approvazione anche unificata perché serenamente destinati a dare certezza alla nostra politica estera e di sicurezza. Mi soffermo invece pochi minuti su un argomento sollevato dal collega Ceccanti nello scorso dibattito di agosto, sul rapporto tra profezia e realismo nell'articolo 11 della nostra Carta costituzionale. Non si tratta di affermare in astratto l'articolo 11 «senza se e senza ma», ma di un atto meditato, legato ad una convinzione profonda: la guerra è impossibile, la pace necessaria. Perché tali affermazioni? Sono illusioni? No, è la Costituzione e il modo in cui si è formata a dircelo: l'articolo 11 sarebbe solo profezia e non anche realismo se non si compone con l'articolo 10 e d'altronde nella logica dossettiana con cui è stato scritto così è. Nulla di strapaesano e locale vi è in questa visione della nostra Carta costituzionale perché essa è coeva alla nascita delle Nazioni Unite nel 1945 a San Francisco: stesso processo costituente. L'articolo 11, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dunque si lega strettamente all'articolo 10 sull'ordinamento internazionale. Nella visione proposta da Dossetti significa il fondamento di uno *ius cogens* precedente al diritto internazionale: gli Stati non stanno insieme nella comunità internazionale in forma pattizia, perché la comunità internazionale, comunità degli degli uomini e delle donne libere, è una comunità originaria che precede gli Stati convenzionalmente dati. In questa comunità di liberi la guerra è rottura della comunità originaria e ogni guerra è guerra civile, perché nega il fondamento stesso dell'essere comunità umana. E questo vale ancor di più per affermare - non solo in via di principio ma nella concretezza delle scelte politiche - la superiorità morale della democrazia contro il terrorismo ed ogni atto violento, anche interno, contro un popolo. È questa visione che ci guida e ci fa dire che ogni vittima (italiana, afgana, irachena, statunitense, spagnola, francese), ogni vittima è nostro fratello o sorella, riconoscendoci nella sua sofferenza. La guerra è il vicolo cieco, il riconoscimento dell'impossibilità di vedere l'altro come simile e sofferente. Uscire da questo vicolo cieco è il compito "regio" della politica. Anche dovrebbe esserlo - il Governo dovrebbe sentirlo - di una politica estera e di sicurezza degna di questo nome. E certo lo si fa partendo dalla situazione reale e dai processi storici. Anche noi lo facciamo, qui ed ora, senza astrarci dal concreto, senza pensare di poterlo fare da soli ma con una inaffondabile volontà di utilizzare il realismo degli articoli 10 e 11 della nostra amatissima Costituzione, affinché sia realizzata anche la profezia felice dell'articolo 11 che ripudia la guerra. È l'utopia in senso giovanneo, ovvero di cosa non realizzata non perché irrealizzabile, ma solo perché mai tentata. Facciamo politica, fate politica: così conquisteremo la pace!

tra manifestanti cosiddetti sabotatori e forze dell'ordine. Lo riferisce un giornale libico. Se andiamo all'articolo 4, comma 23, del decreto missioni scopriamo che 8.297.164 euro sono destinati a garantire «la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani». Voglio sperare che nelle iniziative di oggi, e molto di più, forse, in quelle di domani, quando dovrebbero essere convocate ulteriori manifestazioni, a Tripoli, non venga utilizzato uno di questi euro, che sono stati destinati ormai da due anni a questa parte, al regime del colonnello Gheddafi, che silenzia quotidianamente il dissenso, e lo fa *manu militari*, magari armata coi soldi dei contribuenti italiani. Questo è uno degli esempi che in qualche modo sconfessano l'introduzione del nostro dibattito odierno fatta dal senatore Bettamio, il quale ha detto, senza citare però le percentuali che sono state elencate in maniera puntuale e precisa dal senatore Pegorer, che l'Italia

di cooperazione e sviluppo. Peraltro, queste iniziative di cooperazione e sviluppo, andando a studiare per bene il provvedimento, vengono presentate in modo del tutto

mentre altri soldi sono destinati alla cosiddetta Unione per il Mediterraneo, che non ha fatto niente dal momento della sua fondazione e che, se fosse effettivamente un *forum* dove si prendono in considerazione le realtà del Mediterraneo, magari sarebbe riuscita a fare avere in tempo utile e opportuno un minimo di apprezzamento delle realtà tunisina, egiziana, sudanese

non può (dato che il mandato delle Nazioni Unite non lo prevede) avere niente a che fare con i problemi di politica interna, relativamente alla composizione del Governo. Certo, fortunatamente sono stati destinati degli stanziamenti al tribunale speciale per il Libano, ma questo sicuramente non aiuta a gestire la questione fondamentale, che occorre cioè anteporre la politica alla necessità di dover rispondere alle crisi e alle emergenze con la presenza militare.

di nuovo o non previsto, o che dica cose che la sconfessano come possibile attore politico nella regione. Infatti, se all'indomani delle manifestazioni tunisine auspichiamo che tutto il Medio Oriente assuma il modello Gheddafi per garantire la stabilità,

che verranno affrontate magari in maniera più puntuale quando si arriverà ad esaminare gli emendamenti, perché voglio tornare sulla questione dell'Afghanistan. È stata letta, poco fa, una parte sostanziale della risoluzione adottata nel dicembre scorso dal Parlamento europeo,

redigere i rapporti che provengono da quel Paese. E poi, oltre che lamentarsi di cose su cui ci siamo tutti ampiamente intrattenuti nel passato, si sarebbe arrivati anche alla parte

che per noi resta il problema fondamentale: in quel Paese, fino a quando si manterrà un regime militare di proibizione rispetto all'uso industriale, a fini medici e scientifici, dell'oppio, si continuerà a legalizzare il finanziamento alle reti terroristiche o agli insorgenti. Persistere nella direzione in cui continuate ad andare voi (che senza porvi alcun dubbio rifiutate di fare una minima valutazione dei fallimenti del passato) vuol dire essere conniventi con l'insorgenza.

livello europeo per le missioni ONU e il terzo, dopo la Germania e la Spagna, per le missioni dell'Unione europea. Abbiamo quindi, come è stato sottolineato dai miei colleghi ma anche dai relatori, una grande responsabilità politica, poiché a queste missioni, a cui viene affidato un impegno economico crescente, è anche collegato, avendo 48.000 uomini in campo, a rotazione, lo sviluppo della crescente professionalizzazione dell'esercito italiano e la sua crescente natura interforze. Hanno fatto benissimo il senatore Pegorer, la senatrice Amati e il senatore Del Vecchio a sottolineare il paradosso in cui ci troviamo. Passano i decenni e le legislature; specialmente dal 2001 in poi, sarebbe stato necessario intervenire. Ci troviamo invece sempre qui

e specialmente la natura di queste missioni. Si sta creando infatti quello che viene chiamato il terzo genere delle missioni: azioni militari che però, ciò nondimeno, non sono di guerra. L'ONU e persino la Banca mondiale

non riusciamo ancora a trovare fra noi - il Governo è omissivo in qualche momento e in qualche caso - il nesso fra l'aspetto civile, la cooperazione politica e diplomatica e anche e anche la necessaria azione di forza militare finalizzata al *national building*, al *peacekeeping*, al *peacemaking,* all'attuazione dei piani regionali di ricostruzione e così via. Parlo dell'Afghanistan, e faccio due esempi.

Questo potrebbe essere detto non solo per gli 800 alpini della Taurinense, ma anche per il 2° Reggimento Alpini, che ha fatto la bolla di sicurezza nella valle del Murghab e ha consentito che 6.000 contadini che erano stati scacciati dagli insorgenti e avevano lasciato i loro poverissimi villaggi di montagna ritornassero e trovassero un elemento di continuità civile e di stabilità.

*(FLI)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, con la conversione del decreto-legge oggi in discussione il Governo intende garantire, da una parte, la prosecuzione di alcuni interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e, dall'altra, la proroga della partecipazione delle nostre Forze armate e di polizia a diverse missioni internazionali che si svolgono prevalentemente nell'ambito di territori ad alto rischio o interessati da eventi bellici. Con questo provvedimento si affrontano, dunque, due questioni molto importanti che interessano direttamente tante aree geografiche in tutto il mondo. Situazioni che coinvolgono il nostro personale diplomatico, le nostre Forze armate e di polizia, personale civile operante a tutti i livelli a tutela delle popolazioni locali e degli interessi italiani, dell'Unione europea e della comunità internazionale. Decine di migliaia di italiani sono impegnati a vario titolo: uomini e donne con il loro sacrificio e l'impegno quotidiano rappresentano l'Italia nei contesti internazionali, in scenari di guerra e situazioni di crisi. Uomini e donne, ai quali va il nostro più sentito riconoscimento, che tengono alto il prestigio del nostro Paese e ci consentono di svolgere un ruolo fondamentale a fianco delle più importanti democrazie liberali. Si tratta, signora Presidente, di temi così stringenti e più che mai di attualità, che meriterebbero un'attenzione meditata ed approfondimenti che coinvolgessero il Parlamento ed il Governo insieme in un'azione organica, che non può essere il frutto estemporaneo di provvedimenti di urgenza. di urgenza. Stiamo parlando del ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale e credo che il Parlamento possa e debba interpretare fino in fondo le proprie funzioni, contribuendo in modo propositivo e costruttivo all'azione del Governo in materia di politica estera. Nel corso della mia carriera professionale, quale rappresentante di organismi internazionali, mi sono trovata ad operare in molte delle aree ancora oggi interessate da conflitti o da processi di stabilizzazione e sviluppo. So bene quanto sia importante poter pianificare ed assicurare una presenza ed un sostegno, anche di carattere militare, che coprano un orizzonte temporale sufficientemente ampio, in grado di garantire lo svolgimento e la realizzazione di iniziative di sviluppo che possano godere di un supporto economico adeguato e certo. Per raggiungere tali obiettivi, sarebbe opportuno che il Governo si impegnasse, con il supporto del Parlamento e anche di fronte alla comunità internazionale, in uno sforzo di programmazione che consenta a tutti i soggetti interessati di operare all'interno di un quadro normativo di riferimento chiaro e con risorse economiche assicurate. La via delle proroghe semestrali non è certamente la strada maestra. Per tali ragioni, pur condividendo nel merito il provvedimento in discussione per ciò che riguarda gli interventi in esso previsti, non posso esimermi dal constatare che lo strumento della decretazione d'urgenza non consente di certo gli approfondimenti di cui ho fatto cenno e non garantisce, come in questo caso, una prospettiva temporale adeguata. Al di là delle buone intenzioni, il risultato è che il Parlamento sarà chiamato tra qualche mese ad intervenire nuovamente per prorogare le missioni o per prorogare le missioni o per pianificare ulteriori azioni nelle stesse aree geografiche di cui ci stiamo occupando oggi, e magari anche qualcuna in più. Sappiamo già che le risorse che stiamo per approvare risulteranno insufficienti e che sicuramente il 30 giugno non può rappresentare la data di conclusione delle azioni avviate. Mi auguro, signora Presidente, che nella prossima occasione il Governo operi con sufficiente anticipo in modo da intervenire per tempo, lasciando lo spazio per un corretto confronto parlamentare. Venendo allo specifico del decreto in discussione, per ciò che riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, condivido, come accennato, l'azione del Governo italiano, che conferma l'impegno a partecipare anche finanziariamente almeno fino al 30 giugno, al consolidamento di alcuni programmi di cooperazione in corso in Afghanistan e Pakistan - che io definisco a pioggia - assicurando interventi di carattere sociale, umanitario ed economico, anche attraverso l'impiego delle ONG. L'obiettivo evidente è quello di concorrere alla stabilizzazione delle istituzioni locali e di assistere la popolazione, anche con supporti economici alle imprese in grado di fare ripartire l'economia. Anche per quanto riguarda gli altri Paesi, con le misure previste dall'articolo 2 del decreto, si procede al rifinanziamento di iniziative già avviate e vengono mantenuti gli impegni assunti a livello internazionale. Nello stesso articolo, in sede di discussione parlamentare, sono state inserite alcune piccole ma significative modifiche, di cui vorrei fare cenno. Al comma 1, è stata inserita la previsione di 500.000 euro per assicurare un impegno concreto a favore delle iniziative mirate a prevenire ed eliminare la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Al comma 11, viene stanziato un milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE, istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Considerata la situazione internazionale, specie oggi in alcune aree del Mediterraneo, sono convinta che l'elenco dei Paesi di cui all'articolo 2 è certamente destinato ad allargarsi nelle prossime settimane. Pertanto, la previsione di cui al primo comma, che consente di utilizzare fino al 15 per cento delle risorse disponibili in altre aree di crisi, potrebbe non essere sufficiente -per far fronte alle contingenze internazionali che si determineranno nell'immediato futuro. Per ciò che concerne le missioni di Forze armate e di polizia, segnalo una riduzione cospicua degli interventi nei Balcani, con particolare riferimento alla Bosnia-Erzegovina e al Kosovo. Su questo tema sarebbe opportuno che il Governo decidesse quale politica tenere nell'area. Importanti e significative sono invece le modifiche che riguardano il personale impegnato nelle missioni internazionali. Si interviene non soltanto con disposizioni in materia economica, che pure hanno una loro importanza, specie laddove vengono previste differenze nell'erogazione delle indennità di missione, a seconda dei Paesi in cui opera il personale impegnato, ma, soprattutto, vengono inserite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, norme a tutela della salute e a sostegno delle famiglie, con la previsione di indennizzi nel caso di infermità o patologie tumorali contratte in occasione o a seguito della partecipazione a missioni, con particolare riferimento alle situazioni di personale esposto a particolari fattori di rischio. Insomma, si compie finalmente qualche passo concreto per venire incontro alle esigenze dei militari impegnati in missione, ai fini del riconoscimento delle cause di servizio. In ultimo, sul piano dell'interpretazione giuridica si fa finalmente chiarezza, assicurando la certezza del diritto, anche per quanto riguarda le norme in materia penale. In particolare, attraverso l'applicabilità dell'articolo 4 della legge n. 197 del 2009, viene prevista correttamente la non punibilità dei militari che nel corso delle missioni facciano uso della forza in conformità con le direttive, le regole d'ingaggio e gli ordini legittimamente impartiti.

di rifinanziamento delle missioni internazionali di pace, o per lo meno così erroneamente etichettate - il riferimento all'Afghanistan non è puramente casuale - che, a scadenza semestrale, diviene necessariamente oggetto della nostra analisi e discussione. In questo caso, più precisamente, si assegnano a tali missioni 754.300.000 euro, di cui addirittura 380.770.000 all'Afghanistan. Ho più volte sottolineato, a nome del mio Gruppo, l'assenza di una legge *ad hoc* che disciplini organicamente la materia delle missioni all'estero. A tal proposito, ritengo sia opportuno evidenziare come in Commissione difesa della Camera dei deputati sia inspiegabilmente bloccato, da circa un anno, il disegno di legge n. 2605, presentato dal mio partito e finalizzato a coprire, appunto, tale vuoto legislativo. Ritengo che riprendere questa iniziativa sia una esigenza sempre più impellente e trasversalmente ormai sentita, come confermato anche dalla seduta delle Commissioni riunite 3a e 4a di ieri, alla luce anche del fatto che, negli ultimi dieci anni, l'Unione europea si è affermata come protagonista politica su scala mondiale, assumendosi responsabilità crescenti come attestano le operazioni civili e militari sempre più ambiziose e diversificate, al servizio di un multilateralismo efficace e della pace. A causa di questo maggiore impegno, l'Unione europea ha sicuramente bisogno di sviluppare la propria autonomia strategica mediante una politica estera di sicurezza e di difesa forte ed efficace per affermare le proprie convinzioni nel mondo, per proteggere la sicurezza dei propri cittadini, per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e dei valori democratici, oltre che per salvaguardare la pace in tutto il mondo. In questo scenario, l'Italia, come riporta il resoconto del Ministero della difesa del 13 gennaio 2009, è in termini assoluti l'ottavo Paese fornitore di truppe all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per operazioni di *peacekeeping*, mentre per la stessa esigenza è il primo Paese nell'ambito dell'Unione europea. Ciò vuol dire che migliaia di cittadini italiani appartenenti alle Forze armate e alle forze di polizia sono impegnati all'estero, in missioni al servizio della pace e della sicurezza internazionale. Non è, dunque, più ammissibile l'applicazione di disposizioni inserite di volta in volta nell'ambito di provvedimenti legislativi con cui si dispone un finanziamento per le missioni internazionali. È necessaria una legge di riferimento sul trattamento economico e normativo del personale militare impegnato e sui molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Ecco perché, cari colleghi, ritengo necessario un procedimento legislativo che contenga una serie di disposizioni tese a definire una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali cui partecipa il personale delle Forze armate e delle forze di polizia del nostro Paese. Occorre abbandonare, una volta per tutte, lo strumento della proroga, sintomo, a parere del mio Gruppo, dell'approccio superficiale e approssimativo con il quale si è voluto e si continua a voler affrontare una materia la cui importanza è sotto gli occhi di tutti. Entrando nel merito del provvedimento, riguardo ai fondi destinati precipuamente alla cooperazione e allo sviluppo, occorre evidenziare, anche in questo caso, un dimezzamento delle risorse. Pur essendoci, secondo quanto stabilito nell'articolo 2, comma 1, un ampliamento di 800.000 euro rispetto al precedente finanziamento, la somma stanziata con questa ennesima proroga, 10.500.000 euro, euro, è sensibilmente inferiore alla dotazione di 22.700.000 euro che era stata prevista per il primo semestre del 2010. Sempre da quanto emerge da un'analisi di merito del provvedimento non posso non sottolineare inoltre come, ancora una volta, la metà dei finanziamenti, come precisato in apertura di intervento, siano destinati all'Afghanistan. Nonostante l'impiego di cospicue risorse non si registra però, esimi colleghi, alcun progresso nel processo di pace e stabilizzazione del Paese. Ma mi chiedo, e vi chiedo, cari colleghi: in Afghanistan si può continuare a parlare di missione di pace? Oppure bisogna iniziare ad avere l'onestà morale di pronunciare la parola guerra? Trentasei vite, trentasei nostri ragazzi sono rimasti vittime sul campo di battaglia. Molti altri sono rimasti feriti. Altri ancora sono, per fortuna, scampati agli agguati dei talebani, capaci, in dieci anni di guerra, non solo di difendersi, ma addirittura di riorganizzarsi di fronte ai periodici aumenti di truppe della missione ISAF. Molti civili afgani hanno perduto la vita, soprattutto donne e bambini, la corruzione continua incessantemente a diffondersi in tutto il Paese, la produzione di oppio cresce costantemente, rimanendo la principale fonte di ricchezza del Paese, la condizione delle donne rimane drammatica, nonostante le ragazze abbiano cominciato ad andare a scuola e a frequentare l'università. Non facciamoci abbagliare dal fatto che nel novembre scorso una donna, Maria Bashir, sia stata nominata magistrato. Un evento, questo, sicuramente di portata storica, che però non deve invogliarci a chiudere gli occhi di fronte alle sofferenze quotidiane di molte bambine, date in sposa in tenera età e sistematicamente schiavizzate, picchiate e umiliate dalla poligamia dei mariti. La popolazione civile va sicuramente sostenuta, cari colleghi, rafforzando il supporto ai programmi di sviluppo e di ricostruzione economico sociale messi a punto dalle forze internazionali. In Afghanistan, l'Italia deve aumentare il suo contributo a sostegno della popolazione civile, martoriata da decenni di guerre, e non continuare invece ad avere un ruolo attivo all'interno della missione ISAF, da tutti ormai riconosciuta come una missione di guerra. Il nostro contingente non è però impegnato solo in Afghanistan, ma anche in altri scenari. Mi riferisco alle missioni dislocate in Libano, nei Balcani, in Sudan, in Congo, a Cipro, in Albania, in Georgia, in Iraq e in Somalia, per le quali viene previsto uno stanziamento totale di 373.530.000 euro. euro. Sono angoli del mondo in cui i nostri militari hanno svolto, e continuano a farlo, con grande dedizione e professionalità, una paziente, meticolosa e coraggiosa opera di ricostruzione politica, economica e sociale. Tuttavia, occorre precisare che per tali Paesi, nonostante la complessità delle situazioni in cui versano tali aree, si registra un notevole ridimensionamento delle risorse, soprattutto per quanto riguarda la Somalia dove, a fronte degli 810.944 euro previsti nella precedente proroga, si assegnano 681.198 euro. Una riduzione di risorse ingiustificata, soprattutto alla luce della situazione esistente, peraltro notevolmente complicatasi negli ultimi tempi, sia dal punto di vista politico che umanitario. A fronte di questi tagli ingiustificati assistiamo in questo decreto-legge a degli sprechi e ad una gestione assolutamente non ottimale delle poche risorse in campo. Mi riferisco, colleghi, in particolare a due stanziamenti: il primo in favore del Segretariato permanente dell'Iniziativa adriatico-ionica e il secondo che ha come destinatario il Comitato atlantico italiano. Nell'ambito del progetto di cooperazione nell'area dei Balcani, la Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell'Adriatico, svoltasi ad Ancona nel 2000, ha visto sorgere questa Iniziativa adriatico-ionica i cui membri, oltre all'Italia, sono l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Grecia, la Serbia, il Montenegro e la Slovenia. La IAI non ha organi permanenti ed è destinataria di 300.000 euro. Dalla sua istituzione sono trascorsi ben 11 anni ed è poco chiaro, anche consultando la pagina Internet dedicata, comprendere quale precisa attività svolga tale iniziativa. Non siamo assolutamente in condizioni di verificare l'utilità dell'attività svolta da questa associazione. In assenza di risultati concreti e certi, quindi, diventa molto difficile giustificare una spesa così consistente. Altro stanziamento che desta la nostra curiosità, colleghi, è quello in favore del Comitato atlantico italiano. Tale ente, presieduto eccelsamente dal professore, onorevole La Loggia, svolge una fondamentale, precisa e aggiornata attività di monitoraggio e informazione. È dal sito del Comitato, infatti, che ci siamo resi conto di come le nostre truppe non siano operative nella provincia di Farah, ma siano, piuttosto, ancora stanziate ad Herat. Colleghi, queste sono le assurdità italiane, questi sono gli sprechi italiani, queste sono le vergogne italiane. Con sdegno, mi auguro che almeno quei 250.000 euro previsti per il Comitato, coprano le spese di manutenzione del sito e, quindi, l'aggiornamento delle datatissime mappe e cartine geopolitiche, ferme, nel migliore dei casi, al 2008.

ci tengo a sottolineare e a sottoscrivere quanto siano sacrosante le criticità evidenziate in Commissione dal senatore Torri, che mi aspetto possano essere evidenziate con altrettanta forza ed importanza anche in sede di dichiarazione di voto.

qualitativo e quantitativo da parte del nostro Paese circa l'impegno nelle missioni internazionali,

realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, a significare proprio che la *ratio* delle nostre missioni potrebbe essere sintetizzata nella parola civiltà.

penso che anche in questa occasione, come hanno sottolineato molti colleghi intervenuti prima di me, sia emersa con forza l'esigenza che noi usciamo da questa ordinarietà di discussione del disegno di legge volto le nostre missioni internazionali, per trovarci in un luogo - il Parlamento, su iniziativa del Governo - nel quale aprire una discussione che si faccia carico di osservare, analizzare e quindi, su tali basi, individuare le nuove direzioni di azione, i grandi cambiamenti che sono intervenuti nel frattempo.

che caratterizzano la vita del nostro pianeta, e a me sembra che, almeno negli ultimi due anni, abbiamo evitato di misurarci, di confrontarci e di aprire una discussione su che

soltanto tre, che mi sembrano quelli più rilevanti. Penso innanzitutto ai cambiamenti nel mondo arabo. Siamo passati, all'inizio del nuovo millennio, dalla teoria che bisognava imporre la democrazia con la forza a una situazione nella quale il popolo di quei Paesi si ribella per affermare la democrazia con metodo pacifico. Si tratta di un cambiamento molto rilevante, che induce anch'esso elementi di instabilità che possono interessare la nostra sicurezza, ma di qualità sicuramente inedita rispetto a quelli che abbiamo conosciuto in passato. Il secondo grande cambiamento riguarda la politica degli Stati Uniti d'America, con un Presidente con una grande visione opposta a quella del suo predecessore. In molti, in questi giorni, stanno andando a rileggersi il suo discorso fatto al Cairo appena due anni fa. altro elemento di grande cambiamento è rappresentato dalla crisi finanziaria. Due cose insieme che negli Stati Uniti, ad esempio, provocano un taglio radicale del *budget* per le spese militari, che allontanano gli americani dall'Europa, avvicinandoli di più ai teatri asiatici e mediorientali. Anche questo è un tema nuovo, con il quale dobbiamo assolutamente misurarci.

da questo punto di vista occorre che quello che è accaduto in Tunisia, in Egitto, che sta accadendo in Algeria, e che può accadere in Libia, come è stato ricordato, anche se il Paese è più piccolo, con la popolazione concentrata o distribuita in modo diverso, senza grandi città (tuttavia ci sono movimenti anche lì), ci impone che noi ci ritroviamo a fare un attimo una riflessione su cosa l'Italia pensa rispetto a tutti questi cambiamenti. Questo, perché i Governi cambiano, ma l'Italia resta,

- è realmente quello il posto che occupiamo quando si decide la politica. Questo è l'interrogativo. Segnalo, in conclusione, che il Vice segretario vicario della NATO è sempre stato, da molti anni a questa parte, italiano, mentre si appresta ad essere nominato un americano,

e a questi segnali, che penso non debbano essere trascurati, dobbiamo domandarci se siamo solo truppa nei teatri e consumatori nell'economia, e assolutamente assenti nella politica. Invito il Governo con il suo rappresentante a fare una

*(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, le missioni all'estero sono una componente sempre più importante della politica estera italiana. La partecipazione del personale italiano, sia militare che civile, ad operazioni di gestione delle crisi multinazionali serve gli interessi di sicurezza nazionali, contribuisce a mantenere la credibilità dell'Italia come membro affidabile delle più importanti organizzazioni internazionali di cui fa parte - UE, NATO, ONU - e, inoltre, ne accresce il prestigio internazionale. Al fine di ottenere un miglioramento dell'ottima gestione in corso, propongo di concentrare l'attenzione sulla selezione e sulla gestione politica delle missioni; sull'organizzazione, sull'addestramento del personale e sull'equipaggiamento per le missioni militari di pace; sull'elaborazione di una strategia nazionale per la gestione civile delle crisi; coerenza fra iniziativa politica-diplomatica, azione militare ed aiuti, efficacia, sostenibilità e continuità dell'impegno; sull'entità degli investimenti; sulla proporzionalità tra spese militari e civili; sulla cooperazione civile-militare. Per rendere più aderente il giudizio del Parlamento alla validità della partecipazione alle singole missioni internazionali, appare opportuno impostare una procedura che permetta una valutazione razionale della partecipazione ad un'operazione all'estero, considerando con estrema attenzione i diversi fattori che vado ad indicare: la coerenza della missione con le priorità della nostra politica estera della nostra politica estera e con le politiche delle organizzazioni multilaterali che costituiscono il riferimento dell'Italia in campo internazionale, e parlo sempre di UE, NATO ed ONU. È opportuno indicare inoltre il costo delle missioni in termini di risorse, osservando gli impegni già assunti dall'Italia e mantenendo necessariamente una minima riserva di capacità in caso di emergenza. Attenersi a questi criteri diminuirebbe i rischi di eccessivi sbilanciamenti tra gli obiettivi della missione a cui si è deciso di partecipare e le risorse stesse, sia di personale, sia di mezzi messi in campo. Sarebbe inoltre necessario curare maggiormente la comunicazione con l'opinione pubblica, il cui sostegno è spesso molto importante per la buona riuscita di una missione. Le informazioni dovrebbero essere costanti per tutta la durata della missione. Dovrebbe essere individuato un meccanismo di finanziamento delle missioni più saldo, magari su base annuale e non semestrale, e contestualmente dovrebbero essere rivalutate le Commissioni parlamentari, le uniche idonee alla discussione degli aspetti politici delle missioni, così come proposto da un ordine del giorno accolto dal Governo già due anni fa in occasione di analoga discussione. Sarebbe poi di grande supporto assegnare le risorse - oggi del tutto insufficienti - a disposizione delle Forze armate per le fondamentali attività di addestramento e di mantenimento in perfetta efficienza dei sistemi d'arma e dei mezzi di combattimento e trasporto. Ed infine, ma non meno importante, l'acquisizione degli equipaggiamenti deve rispondere a criteri precisi: essi devono prestarsi ad un utilizzo mirato in modo da premiare il rapporto costo-efficacia per ottenere la migliore protezione possibile del personale; nel contempo, signora Presidente, si deve garantire ai pacchetti di impiego costituiti *ad hoc* la disponibilità sicura di sistemi d'arma e di acquisizione obiettivi per garantirne la migliore capacità operativa. *(Applausi dal

dell'Aula al provvedimento in esame, e quindi, nella sostanza, alla presenza italiana in molti teatri internazionali attraverso le missioni militari e l'azione di cooperazione allo sviluppo, oggetto di una parte del provvedimento

ci troviamo a prorogare gli impegni internazionali del nostro Paese, si devono rilevare alcune

in una contingenza economica e in una sorta di crisi complessiva che non facilita sicuramente il reperimento

nell'ambito della cooperazione lo sviluppo, che costituiscono parte del provvedimento in oggetto. Il Parlamento ha

in questa direzione; ma ha anche il dovere, altrettanto importante, di individuare possibilità concrete e reali perché detti auspici e indicazioni non si limitino a luoghi a luoghi comuni, a petizioni di principio che difficilmente possono trovare una qualche forma di realizzazione. Si deve sicuramente

di disporre di un quadro di riferimento normativo certo, definito e che travalichi la temporaneità dei decreti che ormai

concorde sulla possibilità di intensificare i tentativi per raggiungere uno strumento che possa soddisfare alcune esigenze che sono state in questa sede ricordate da più parti; ma bisogna essere realisti: non si può pensare di definire tutto quanto è contenuto in questi decreti periodici perché, come dicevamo all'inizio, la parte riferita agli impegni finanziari difficilmente potrà trovare una connotazione diversa per l'attuale situazione e, d'altra parte, così è stato sostanzialmente da quando questi decreti hanno cominciato ad essere

temporale è stato di un anno o di tre mesi, la cadenza dei sei mesi è stata mantenuta, non soltanto nelle tre legislature che si sono succedute, ma dai vari Governi di pur differente colore che

può trovare adeguata normazione nell'ambito dell'emanando - auspichiamo - codice penale militare per le missioni internazionali. gli intervenuti hanno sottolineato la grande rilevanza, sotto più aspetti, degli interventi del nostro Paese nei vari contesti. Certamente, alcune critiche che fanno alcune critiche che fanno riferimento a parti specifiche del provvedimento hanno un sapore non sempre conforme allo spirito generale. non credo, senatore Perduca, che le risorse, peraltro abbastanza limitate, riferite alla manutenzione delle motovedette in uso per l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, cedute temporaneamente dall'Italia alla Libia con personale parzialmente italiano, possano essere utilizzate a fini diversi se non quelli per i quali sono state previste. Escludo che possano essere utilizzate per il contrasto delle insurrezioni interne o delle attività di protesta democratica. inoltre aver udito qualche considerazione decisamente superficiale - me lo consenta - in ordine alle risorse destinate all'*intelligence* che, a suo dire, sarebbe stato meglio destinare a qualcos'altro,

di risorse per l'azione di *intelligence*, si deve sempre ricordare un luogo comune, ma anche un'evidenza, e delle attività di *intelligence* difficilmente si possono verificare i risultati positivi: infatti, anche quando, grazie a delle informazioni che spesso, ma non sempre, purtroppo, si riescono ad ad avere in anticipo riguardo a minacce e pericoli che possono coinvolgere i nostri contingenti, molti attentati e azioni offensive sono stati scongiurati e molte vite sono state risparmiate, questo non ha potuto, e non può, costituire oggetto di grande manifestazione pubblica e deve rimanere nell'ambito di quella riservatezza che è propria dell'azione di*intelligence.* È ingeneroso dire che l'azione di *intelligence* dei nostri servizi non abbia contribuito efficacemente alla protezione dei nostri dei nostri contingenti. Comunque, è di tutta evidenza che per quanto in tutti i settori - e questo non vale soltanto per l'*intelligence*, ma evidentemente anche per la dotazione dei mezzi, per le corazzature e gli strumenti di individuazione preventiva - tutto possa essere migliorato e perfezionato, non ci sarà mai la possibilità di garantire una sicurezza assoluta e un'eliminazione totale dei pericoli, proprio perché, come tutti hanno ribadito, nell'ambito in particolare dello scenario afgano, la situazione è quella in cui non si può parlare di un conflitto in senso tradizionale, ma certamente di una situazione in cui, come è a tutti noto e

non può nemmeno sottacersi quanto è stato ricordato in più interventi. Ringrazio in particolare la senatrice Negri che ha fatto un giusto ed opportuno elenco delle azioni positive di carattere non strettamente militare, ma che non possono che essere garantite dallo strumento militare riguardo allo scenario afgano, riferendo delle operazioni compiute dagli alpini della Brigata Taurinense a titolo esemplificativo. Infatti, le azioni che lei ha ricordato ed elencato sono le stesse che quotidianamente ogni reparto dei contingenti militari italiani, in quello scenario in particolare, compie, proprio perché lo strumento militare è quello che consente la creazione di quegli ambiti di sicurezza, le famose bolle, che innanzitutto restituiscono alla libera frequenza e alla libera disponibilità delle popolazioni porzioni di territorio sempre più vaste che erano invece loro state sottratte e in cui la loro presenza era stata interdetta proprio dall'azione degli esponenti talebani e delle milizie talebane. E se questo è vero, ed è opportuno ricordarlo nelle occasioni in cui svolgiamo questi dibattiti, d'altra parte, però, non si può poi far finta che questo non sia e non comprendere che, anche attraverso questa forma di lettura, si individui

è una fascia intermedia molto ampia, fatta di azioni finalizzate alla ricostruzione, alla riproposizione di condizioni di sicurezza, ma anche di di convivenza civile che vengono svolte dagli operatori militari e che quindi devono essere considerate nella loro reale portata anche nell'ambito delle finalità complessive, che sono quelle, in molti casi, di creare le condizioni di pace, di ricreare le condizioni di pace, di costruire la pace. È troppe volte misconosciuto il valore che alle alle stesse definizioni viene dato quando si parla genericamente, e forse sbagliando, di missioni di pace. No: sono situazioni molto diverse, anche quelle presenti nei vari contesti in cui sono tante - 30 e oltre - missioni elencate in questo, come negli altri provvedimenti precedenti. Ancora una volta, nemmeno si può può misconoscere, modificare la reale portata del sempre citato articolo 11 della Costituzione

che lo Stato, in questo caso italiano, svolga delle operazioni militari e che sono per certi versi non soltanto puramente difensive, ma in determinati ambiti, anche preventive riguardo alle situazioni di pericolo: rifiuta la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali, cosa ovviamente molto diversa rispetto a ciò che molte volte viene invocato, anche perché, se così non fosse, ovviamente tutte queste missioni e tutti questi provvedimenti che le riguardano sarebbero contrari alla Costituzione, cosa che, viceversa,

ma adeguate a questi rilevanti impegni che vengono richiesti. Anche in riferimento a tale aspetto, è necessario che si facciano i dibattiti, che si affrontino le questioni generali, che si valuti che cosa si ritiene di fare in ordine al futuro, al prossimo decennio delle Forze armate e agli interventi italiani nei vari contesti internazionali, ma cominciamo già da queste occasioni ad esprimere valutazioni in ordine alla questione fondamentale che certamente potrebbe e dovrebbe costituire l'oggetto di questi dibattiti: il Parlamento e le forze politiche ritengono adeguato l'impegno italiano, quantitativo e qualitativo, nell'ambito delle missioni internazionali, dei vari scenari e della presenza nella cooperazione fra gli Stati

quanto riguarda la sicurezza interna, dai confini naturali e tradizionali ad ambiti molto più lontani, da cui peraltro, come è stato più volte dimostrato nel corso di questo decennio e di quello precedente, sono partite azioni offensive che hanno coinvolto e colpito la sicurezza dei cittadini, europei di molti Stati, oltre che ovviamente quella dei cittadini e dei civili degli Stati Uniti d'America, a cominciare dall'attentato alle Torri Gemelle e da quelli coevi. Credo che questo sia l'oggetto principale su cui ci dobbiamo confrontare: se si ritiene che l'impegno italiano sia idoneo e conforme a quanto il Parlamento auspica e ritiene, allora,di conseguenza, si deve discutere se l'impegno militare è conforme a questi impegni e a questa volontà di presenza italiana. È su questo che deve svolgersi un confronto corretto. Certamente, si devono ritrovare le occasioni per valutare i grandi cambiamenti di cui parlava il senatore Cabras, ma quei cambiamenti in qualche modo prescindono dalla prosecuzione delle missioni di cui stiamo parlando nell'ambito della conversione di questo provvedimento. Sono certamente situazioni di scenario che il Parlamento non può non considerare, ma che non credo possano fare venir meno quell'importanza, quella determinazione e quella considerazione positiva che sostanzialmente tutti hanno confronti di tale impegno, che deve trovare anche nel voto finale e nella conferma di quella larga condivisione quella solidarietà e quel senso di vicinanza concreto che da parte delle Assemblee parlamentari viene a tutti i nostri militari, a tutte le donne e gli uomini con le stellette che sono impegnati non soltanto all'estero ma anche in Patria affinché quelle missioni possano portare ad esiti favorevoli.

a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. La legge è stata infatti approvata dal Senato della Repubblica il 14 febbraio di dieci anni era or sono. Si è trattato di un traguardo importante, e non solamente per gli appartenenti alla comunità linguistica slovena, perché con essa si è data attuazione agli articoli della Costituzione ed al riconoscimento storico di tutti gli appartenenti alla comunità slovena, indipendentemente dalla provincia di residenza (cioè Trieste, Gorizia e Udine). È stato un avvenimento importante anche per l'intera comunità locale, visto che la legge, improntata alla gradualità, alla condivisione, alla partecipazione, ha contribuito ai processi di integrazione, di convivenza, come anche - penso di poterlo dire - a creare un clima disteso, un clima positivo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica italiana, come abbiamo potuto constatare recentemente con la visita del presidente Türk a Roma. Colgo questa occasione però anche per sottolineare che alcune parti della legge sono tuttora inattuate. Vi ho fatto cenno molte volte negli interventi svolti in Aula ed in diverse interrogazioni. solo alcuni esempi: l'istituzione della sezione slovena presso il conservatorio di musica «Giuseppe Tartini», la corretta scrittura dei nomi e cognomi, la la restituzione di tre beni immobili citati nella legge. Chiedo a questo proposito al Governo, ai singoli Ministri, ai loro uffici periferici, agli enti locali di impegnarsi affinché tutte le parti della legge vengano applicate ed attuate e sia così

previsto al comma 9 dello stesso articolo: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa».

È una norma scritta sotto diretta dettatura dei banchieri per umiliare, ancora una volta, i giudici della Suprema corte e i sacrosanti diritti di milioni di consumatori e utenti dei servizi bancari, massacrati da una cricca

che Governi, di destra e di sinistra, in ossequio ai *desiderata* dei banchieri, tentano di cancellare le sentenze della Suprema magistratura, costate lacrime e sangue. Anche il senatore Legnini, che voglio ringraziare, ha sollevato nel suo intervento l'estraneità della norma salvabanche al decreto milleproroghe, arrivata all'ultimo minuto proprio per non essere esaminata dalle Commissioni riunite 1a e 5a Per questo, lascio agli atti del Senato l'annuncio di un'impugnativa delle norme approvate, in particolare di questo colpo di spugna sulla prescrizione, con ricorso nei tribunali, per sollevare eccezione di legittimità costituzionale di norme salvabanche inserite all'ultimo secondo per impedire che i senatori potessero discuterle e opporsi, sottratte quindi al dibattito per cancellare i sacrosanti diritti sanciti dai giudici delle sezioni unite civili della Cassazione. La

Volevo ringraziare il sottosegretario Scotti per aver risposto a queste due interrogazioni, ma ancor di più la Farnesina per aver acconsentito ad una missione, organizzata in poche ore, alla quale hanno partecipato anche gli onorevoli Mecacci e Pannella,

insieme anche al sottosegretario Scotti - saranno presenti al 39° congresso del Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito che si terrà a Chianciano e al quale colgo l'occasione per invitare tutti i presenti a partecipare, di promozione e di difesa dei diritti umani. Entrambe le risposte del sottosegretario Scotti ricordano che la Farnesina continua ad essere impegnata, a livello bilaterale e nel quadro europeo, per la promozione dei diritti umani in Mauritania, dove esiste ancora la schiavitù. In particolare, auspico che l'impegno italiano in quella parte del mondo si concentri sulla discriminazione razziale - perché molto spesso, anzi nella stragrande maggioranza dei casi,